da parte del presidente del Consiglio Conte sugli esiti della Conferenza sulla Libia che si è chiusa ieri. Siamo davvero preoccupati per quanto è successo: la Conferenza si è chiusa con un nulla di fatto, senza alcun documento. Vorremmo comprendere meglio gli esiti, declamati solo come auspici rispetto al futuro della Libia, un Paese che a noi interessa

del Mediterraneo hanno lasciato la Conferenza anzitempo. C’è stato poi il balletto degli ospiti, con Haftar che è arrivato a Palermo, ma non ha partecipato alla Conferenza. Su un dossier così importante, su cui era stata stata alzata la posta in gioco ed erano state elevate le aspettative, noi ci aspettiamo a brevissimo un intervento del presidente Conte, che venga a riferire in Senato sugli esiti della Conferenza, ma soprattutto sui sui prossimi appuntamenti che dovranno vedere l’Italia protagonista in Libia, affinché arrivino risposte chiare sul versante delle possibili elezioni e del coinvolgimento dei principali attori. Ad oggi non sappiamo nulla di tutto questo e quindi pensiamo che sia opportuno - questo è il motivo per cui ci sarà una richiesta netta da parte del Gruppo del Partito Democratico - che il Presidente

recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Signor Presidente, onorevoli senatori, membri del Governo, prima di entrare nel merito del provvedimento che giunge oggi all’esame di questa Assemblea, vorrei rivolgere un sentito ringraziamento ai Presidenti e a tutti i senatori delle Commissioni riunite, alle forze di maggioranza, al mio Gruppo, al senatore Romeo, per avermi consentito di svolgere, in quanto senatore ligure, il ruolo di relatore per l’8[a] Commissione, di cui non sono un componente titolare. Allo stesso modo ringrazio il senatore Pepe, che ho sostituito nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione lavori pubblici. Mi soffermerò pertanto sulle norme del decreto-legge di cui si propone la conversione che riguardano gli interventi messi a punto dal Governo per fornire il necessario sostegno al territorio e alla popolazione di Genova, così profondamente colpiti dal crollo del viadotto Polcevera, per favorire la ripresa economica di quei territori, nonché per innalzare, più in generale, il livello di sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è giunto all’esame del Senato con numerose integrazioni e riconosciuti miglioramenti dopo l’approfondito esame svolto presso la Camera dei deputati, passato anche attraverso l’ascolto dei rappresentanti istituzionali dei territori coinvolti del mondo del lavoro, delle imprese e della società civile. Il lavoro svolto dal relatore, 1’onorevole Flavio Di Muro per la parte di competenza dell’8[a] Commissione, ha appunto consentito di vedere riconosciute tutte le esigenze all’interno del decreto-legge oggi in approvazione, mostrando la sensibilità del Governo in merito alla tragedia che ha colpito Genova e i suoi abitanti. Mi si permetta altresì di ringraziare il Governo ed in particolare il vice ministro Rixi che da ligure e genovese ha saputo far vedere riconosciute le esigenze di Genova e dei genovesi in questo provvedimento, consentendo alla città di poter guardare con fiducia al futuro in termini di rilancio e competitività. La necessità di consentire l’avvio immediato delle attività di ricostruzione e di aiuto alla popolazione, impongono ora di procedere al più presto con la conversione del decreto-legge, per rispettare i termini costituzionali ma soprattutto per accelerare l’entrata in vigore delle norme introdotte alla Camera: penso in particolare alle misure per gli sfollati. Mi preme ora ringraziare il Governo per l’apertura dimostrata durante l’esame nelle Commissioni riunite, mediante l’accoglimento della maggior parte degli ordini del giorno presentati sia dalle forze di maggioranza che di opposizione: degli 89 ordini del giorno esaminati, infatti, il Governo ne ha accolti 55 nel testo dei proponenti, 21 in un testo riformulato dai presentatori e infine ne ha accolto uno come raccomandazione. Quanto al testo del provvedimento, il Capo I contiene le norme su Genova. In particolare, l’articolo 1 disciplina l’istituzione e i poteri del commissario straordinario per la ricostruzione,

- operi in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo, oltre al rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Diverse disposizioni regolano poi i rapporti tra il commissario straordinario e la società Autostrade per l’Italia SpA. In particolare, è stabilito che il concessionario del tratto autostradale, alla data dell’evento, sia tenuto a far fronte alle spese di ricostruzione dell’infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario. In caso di omesso versamento, il commissario potrà procedere all’individuazione di un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere. A garanzia dell’immediata attivazione del meccanismo di anticipazione, per assicurare il celere avvio delle attività del commissario, è comunque autorizzata la spesa di 30 milioni annui dal 2018 al 2029. Il commissario straordinario può procedere ad affidare, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario a soggetti diversi dal concessionario del tratto autostradale e da società o soggetti da quest’ultimo controllati

L’esclusione della società Autostrade dalla realizzazione delle attività di ricostruzione è motivata con l’eventualità che il concessionario sia responsabile, in relazione all’evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio. L’articolo 1-bis, finalizzato alla tutela del diritto all’abitazione, disciplina la procedura per le cessioni volontarie e gli eventuali espropri delle unità immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero emanate in seguito al crollo del ponte Morandi, con la previsione della corresponsione di un’indennità ai proprietari e agli usufruttuari, posta a carico del concessionario del tratto autostradale. L’articolo 1-ter introduce misure specifiche per l’esecuzione delle attività di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi e per la verifica e messa in sicurezza, da parte delle concessionarie autostradali, di tutte le infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, con particolare riguardo a ponti, viadotti e cavalcavia. Per fronteggiare le necessità conseguenti al crollo del ponte Morandi, l’articolo 2 autorizza l’assunzione di personale da parte degli enti territoriali e dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale.

L’articolo 3 contiene una serie di agevolazioni fiscali per gli immobili che a seguito del crollo del ponte Morandi hanno subìto danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero. È stata inoltre introdotta la possibilità di prevedere l’esenzione dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia. Con l’articolo 4 sono riconosciuti benefici economici alle imprese e ai liberi professionisti, con sede operativa all’interno della zona danneggiata, che abbiano subìto un decremento del fatturato, mentre con l’articolo 4-bis, in analogia con quanto stabilito per le famiglie all’articolo 1-bis del decretolegge, sono introdotti indennizzi per la cessione volontaria o l’esproprio degli immobili che ospitano le imprese che abbiano subito danni. Anche in questo caso, gli oneri sono posti a carico del concessionario autostradale. La medesima previsione vale anche per il ristoro della perdita e dei danni subiti dalle attrezzature e dai materiali aziendali. In deroga alle disposizioni generali in materia di ammortizzatori sociali, l’articolo 4-ter dispone che venga concessa ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, penalizzati nell’attività lavorativa, un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale. Un’indennità una tantum è poi riconosciuta ai titolari di rapporti di collaborazione coordi- nata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi che abbiano dovuto sospendere l’attività a seguito del crollo. L’articolo 5 prevede stanziamenti per il finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi, per l’efficientamento del trasporto pubblico regionale e locale, per l’integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nel territorio della città metropolitana di Genova. Sono poi destinati 20 milioni per il 2019 e per il rinnovo del parco mezzi utilizzati, con priorità per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno. Con riferimento all’autotrasporto, sono stanziati 20 milioni di euro per il 2018 per il ristoro delle maggiori spese affrontate in conseguenza del crollo del ponte Morandi. Per la realizzazione di opere viarie di collegamento o comunque inerenti la mobilità sono attribuiti 5 milioni di euro al Comune di Genova. che, con riferimento alle opere individuate come itinerari di viabilità alternativa, il commissario delegato possa autorizzare varianti in corso di esecuzione in deroga all’articolo 106 del codice dei contratti pubblici. L’articolo 6, al fine di garantire l’ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di sovraintendere alla progettazione e alla realizzazione, in via d’urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie.

Con l’articolo 7, al fine di superare l’emergenza e favorire la ripresa delle attività economiche, viene istituita la «Zona Logistica Speciale - Porto e Retroporto di Genova», con la previsione dell’applicazione di procedure semplificate per le imprese che avviino un programma di attività imprenditoriali o di investimenti nei territori in essa ricompresi. Sono poi previsti contributi finalizzati a sostenere il trasferimento di una quota di trasporto merci da gomma ad altre modalità, con particolare riferimento al trasporto ferroviario, con la previsione anche di compensazioni per il concessionario del servizio di trasporto ferroviario. L’articolo 8 istituisce, nell’ambito del territorio della Città metropolitana di Genova, una zona franca urbana, con la concessione di una serie di agevolazioni fiscali per le imprese ivi stabilite. L’articolo 9 incrementa, per gli anni 2018 e 2019, la quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti riconosciuta ai porti ricadenti nell’ambito dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, destinando inoltre a tale Autorità un contributo aggiuntivo di 4,2 milioni di euro per il 2018. L’articolo 9-bis dispone che il commissario adotti un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura dell’Autorità di sistema portuale con l’applicazione delle deroghe già definite dall’articolo 1 del decreto-legge in esame. del decreto-legge in esame. L’articolo 9-ter, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso il porto di Genova, proroga di cinque anni l’autorizzazione attualmente in corso per l’esercizio dell’attività di fornitura di lavoro temporaneo e prevede la possibilità che venga corrisposto

Il capo II contiene disposizioni per la sicu- rezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti. L’articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture l’articolo 13 si procede all’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), il cui sviluppo risponde alla necessità di garantire una costante verifica dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni ricavate dal Sistema di monitoraggio dinamico per

Go- verno, onorevoli colleghi, mi associo ai ringraziamenti del collega Ripamonti alle Presidenze e agli Uffici delle Commissioni riunite 8[a] e 13[a], che hanno lavorato con grande capacità,

Svolgerò la relazione per quanto riguarda i capi dal III in poi di un decreto-legge che reca misure importanti per l’enorme tragedia che ha colpito Genova e la Liguria, ma anche per tutto il Paese, perché Genova è una città fondamentale per il

Mi riferisco, quindi, agli interventi per il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia, per un combinato disposto di 20 articoli (quindi non soltanto uno, come una narrazione fuorviante sta cercando di far passare). Si tratta di 20 articoli che consentono, innanzitutto, di definire l’ambito di applicazione del commissario straordinario, che modulano, rimodulano e ampliano le funzioni del commissario. L’articolo 19 incrementa di 60 milioni di euro la contabilità speciale per il commissario. Vi sono interventi che riguardano la ricostruzione pubblica e la ricostruzione privata, i criteri e le modalità generali per la concessione di contributi per la ricostruzione privata; interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti; interventi di immediata esecuzione e le procedure per le concessioni ed erogazioni dei contributi. Si tratta di un terremoto che forse

Ha distrutto case, vite, aziende, tessuto economico e produttivo, turismo; ha portato via due persone, quindi due famiglie e interi nuclei familiari distrutti da una tragedia.

Nessuno ricorda, però, che quel terremoto ha avuto una caratteristica quasi unica nei terremoti italiani, ossia quella di avere un epicentro molto superficiale,

Ischia, vi sono ovviamente i fondi per la ricostruzione pubblica, la definizione dei soggetti attuatori, norme per la legalità e la trasparenza, la qualificazione degli operatori economici

e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. C’è la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e gli interventi volti alla ripresa economica. C’è anche il famigerato articolo 25, che non è un condono edilizio. Non lo è, perché non esiste un’apertura di termini per la presentazione di nuove domande. Non lo è, perché nessuno che non aveva diritto ieri di avere la casa condonata ce l’avrà oggi. (Applausi perché la procedura che si segue è l’unica disponibile nella legislazione vigente, cioè quella della legge n. 47 del 1985: l’unico condono che ha definito le procedure per il rilascio delle pratiche. Quindi, se avessimo fatto riferimento alle leggi nn. 724 e 326 rispettivamente del 1994 o del 2003, non avremmo avuto la procedura.

su cosa potrebbe accadere se non ci fosse l’articolo 25: quelle case, che sono danneggiate e alcune di loro crollate, sarebbero fuori dalla procedura di accesso ai contributi. Ricordo, peraltro, che nessuna parte di volume edificato senza concessione potrà essere ammesso a contributo. Quindi, le parti di volume edificato in modo abusivo e condonate ai sensi della legge n. 47 del 1985, della legge del 1994 e della legge del 2003, con le procedure che impostiamo oggi come accelerazione, avranno la possibilità di essere condonate secondo la domanda fatta quindici o trent’anni fa, ma non avranno ovviamente accesso al contributo per la parte di volume sanato. Ribadisco: che cosa succede se non c’è l’articolo 25? Quelle case hanno comunque una domanda pendente

la possibilità di intervenire per sistemarle e recuperare i danni prodotti dal terremoto, non solo continueranno ad avere una casa abusiva, non solo continueranno a viverci dentro, ma avranno una casa indebolita dai danni del terremoto. Questo è il vero pericolo per questo che chiediamo un’accelerazione delle procedure per dichiarare illegittime le domande che non sono in regola con il condono di appartenenza (quindi i condoni del 1985, del 1994

provvede a rimodulare le misure per l’accelerazione del processo di ricostruzione e le funzioni del commissario. Si provvede a garantire l’impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate dagli eventi sismici. inoltre ad ampliare quelle maglie che, con i guanti bianchi e con il contributo di tutte le forze politiche, avevamo reso molto strette per piccole difformità,

ricostruzione o riparazione dell’edificio si sana anche la parte realizzata eventualmente ai sensi dei piani casa regionali e, anche in questo caso, sul volume così sanato non si applica il contributo. Vi sono altri due elementi che voglio segnalare. Il primo concerne l’articolo 44, sul trattamento straordinario integrazione salariale per le imprese in crisi. reinserito nell’ordinamento la Cassa integrazione guadagni straordinaria per le aziende in crisi che hanno una prospettiva è, a mio giudizio, un valore di cui anche il centrosinistra dovrebbe essere contento. Cerchiamo, in questo modo, di dare qualche garanzia in più ai lavoratori delle aziende, che attraversano una crisi ma hanno una prospettiva e che per problemi di liquidità non riescono a garantire un’attività produttiva. Quindi, grazie a tale misura,

il 41. Oggi, dopo più di vent’anni di spargimento di fanghi, senza che vi sia stato mai nessun limite ai contenuti nocivi di quei fanghi, anche riguardo agli idrocarburi e agli altri inquinanti, ci rendiamo conto che questo è un problema per la nostra salute. Noi ce ne rendiamo conto, come ci rendiamo conto del fatto che è un problema riguardante la nostra salute

di mare, o in altri canali le acque depurate prive del fango. Questo è quanto succede se non si interviene con la nuova norma emergenziale. Io non sto a ripetere le considerazioni che abbiamo già fatto su questa norma in Commissione. Dico solo che c’è un impegno del Governo a normare in modo definitivo, chiaro e certo il problema dell’utilizzo dei fanghi in agricoltura. Io sono convinto che il nostro Ministro dell’ambiente, che è un generale dei carabinieri che di questi temi si è occupato per tutta la vita, perseguitando chi con i rifiuti faceva affari, saprà emanare in tempi rapidissimi un decreto che normerà in via definitiva questo problema. Oggi, però, c’è un’emergenza, che trattiamo con senso di responsabilità, grande capacità e competenza

si adegua) il clima del monocameralismo di fatto. Si blindano i provvedimenti: è stata approvato alla Camera e non volete che si modifichi al Senato. Eppure, ci sarebbe molto da modificare. Il buon lavoro dei colleghi, anche dei relatori, ai quali do atto dell’impegno, avrebbe potuto produrre effetti positivi ed importanti. Ma voi non volete cambiare nulla. Vi avevamo chiesto di togliere di mezzo il condono ad Ischia. Collega Patuanelli, il problema non è l’emergenza Ischia. Il problema è che il condono non è un’emergenza. È molto semplice: il condono non è un’emergenza per nessuno e, a maggior ragione, non lo è per noi. Togliete i fanghi di depurazione: e tornerò

che portano cose mefitiche, e non solo perché si parla di fanghi. Il ministro Costa, citato un attimo fa dal collega Patuanelli, ha detto:

in televisione ho sentito il procuratore capo Cozzi, la cui autorevolezza mi pare sia indiscutibile e indiscussa, il quale, rispetto alle proteste del commissario perché il cantiere è ancora sotto sequestro e non si possono non si possono avviare le azioni di demolizione, ha detto che dovrebbero ringraziarlo perché se gli restituisse il cantiere non saprebbero cosa fare. Il condono non risolve neanche il tema della demolizione; non si sa neppure chi deve metterci mano e come. La strada maestra era non fare propaganda, non cercare colpevoli in forze politiche che nessuna responsabilità avevano. La strada maestra era quella di un vecchio adagio: chi rompe, paga. Penso anch’io che la società Autostrade per l’Italia abbia delle responsabilità; la si obbligava a demolire e a realizzare il ponte, e poi ci si rifaceva su di essa in tutti i modi, anche con la revoca che avete invocato e che non avete fatto, cosicché, come tutte le vostre parole di propaganda, si rimane a mezza strada, senza sapere

fermo. Il meccanismo che avete scritto nel decreto-legge, secondo cui paga Aspi, e, se non paga Aspi, un finanziatore si rifarà su Aspi, mi sembra molto complesso: auguri, auguri al nostro Paese, ma soprattutto ai cittadini genovesi che, attraverso queste vostre complicazioni, rischiano di non vedere mai la strada ricostruita. D’altra parte, non avete cultura in materia infrastrutturale: Toninelli un giorno realizza il tunnel del Brennero; in un altro fa la radiografia di un viadotto a vista; in un altro ancora dice che si potrà mangiare sotto un ponte autostradale. Nel frattempo, tutto fermo. Accogliete almeno i nostri emendamenti di buonsenso, che danno una risposta immediata ai cittadini di Genova, che non hanno più voglia di applaudire i rappresentanti di questo Governo. PRESIDENTE. Senatore Margiotta, mi perdoni se la interrompo. Colleghi, il livello del brusio è insopportabile. Se non c’è rispetto per il relatore, chiedo almeno il rispetto per i colleghi che vogliono ascoltare il relatore. Vi ringrazio.

ma la ratio per la quale non si approva neppure un ordine del giorno che dice che bisogna procedere nei lavori del Terzo valico è assolutamente incognita. Anzi, è nota: non avete voluto approvarlo per evitare problemi tra le due forze che sorreggono questo Governo, di cui una pensa che il Terzo valico - vero, vice ministro Rixi? - vada realizzato, e l’altra ancora non ha deciso e aspetta una fantomatica analisi costi-benefici, su cui tornerò durante la replica, che non può dare alcuna risposta, come ha detto un esperto della materia, lo stesso esperto che avete nominato. I costi, infatti, sono certi, almeno alla fine della costruzione dell’opera; i benefici derivano da una scelta politica, perché quel che è beneficio per una forza politica non lo è per un’altra. Infatti cosa ha detto, in

Peraltro, l’analisi costi-benefici su un’opera che ha uno stato di avanzamento al 40 per cento è abbastanza risibile. Torno al condono. Durante il terremoto di Ischia è caduta una sola palazzina, che aveva sopraelevato un piano, mettendo a rischio l’incolumità della famiglia con figli e dei terzi che vi abitavano. I condoni sono fatti anche di questo, mica soltanto delle ringhiere e dei balconi o delle tettoie

i comportamenti dei colleghi del MoVimento 5 Stelle, quando si dipingevano le mani nere a significare che il petrolio inquina. Benissimo:

non contenti, alla Camera avete aumentato i limiti di concentrazione del cromo, dell’arsenico, del toluene e di altro in fanghi che vanno a finire anche in terreni in cui si coltivano colture alimentari, dove viene coltivato ciò che arriva sulle nostre tavole. È evidente che abbiamo appoggiato e appoggeremo l’emendamento Martelli, come quello a prima firma De Bonis e di una decina di altri componenti del Gruppo MoVimento 5 Stelle. Loro sono coerenti con quanto il vostro partito ha detto per cinque anni;

Ma torneremo sul merito di ciascuno di questi emendamenti nel corso della discussione, augurandoci sempre che ci sia un sussulto di dignità. Ieri è accaduta una cosa importante, è volgare aver derubricato a questioni personali, perché riguarda colleghi seri e autorevoli, che hanno dimostrato di esserlo nella loro vita privata e in quella parlamentare.

ma ci sarà sempre qualcuno che avrà autonomia, coscienza e libertà di azione e di pensiero: queste persone vi inchioderanno alle vostre responsabilità.

Presidente, è che in tre mesi di lavoro questo Governo ha parlato di Genova, ma non ha fatto praticamente nulla. Quello che avrebbe dovuto essere il provvedimento centrale, in realtà, è stato deprivato di qualsiasi efficienza ed efficacia a favore dello sviluppo di Genova.

perché l’intervento per cui si fa domanda è totalmente all’interno, con il duplice concetto di conformità, di quanto previsto dalla programmazione urbanistica comunale.

L’ultima questione, Presidente, come spiegato bene dal relatore Margiotta, concerne lo spandimento dei fanghi. Il tema è serio; noi non facciamo demagogia e non cambiamo le nostre casacche, bandierine e comportamenti a seconda che siamo al Governo o all’opposizione, come fanno le attuali forze di maggioranza. La questione dei fanghi è un tema vero, ma è del tutto sbagliato inserirlo nel provvedimento al nostro esame. I fanghi hanno bisogno di un provvedimento organico. Siccome la legge non consente nei mesi invernali lo spandimento dei fanghi nei campi da dicembre a febbraio, c’è tutto il tempo di

provvedimento al nostro esame doveva essere il decreto delle emergenze, se di emergenze vogliamo parlare, oltre a Genova, che è l’emergenza madre da cui parte il provvedimento e per la quale dobbiamo dare tutto il nostro contributo e sostegno, c’è un’emergenza che è nata nelle nostre città, nei nostri territori, in undici Regioni che nelle settimane trascorse hanno chiesto lo stato di emergenza. Voi avete tolto, avete ucciso e negato Casa Italia e Italia sicura, che erano le unità di missione e i dipartimenti che davano reale risposta all’emergenza sismica ed idrogeologica.

Per voi l’emergenza è il condono e non sostenere le comunità gravemente colpite dal disastro ambientale delle scorse settimane? Abbiate la decenza di fare un provvedimento ad hoc perché i territori aspettano risposte immediate.

Presidente, onorevoli colleghi, cosa ac- comuna le tematiche trattate nel decreto Genova? Le emergenze, problemi da risolvere prima possibile. Ci si deve chiedere se un disastro di questa entità fosse evitabile e di chi sono le responsabilità, in modo da non rischiare di subirne di simili. La cosa più semplice è associare il disastro alla mancata manutenzione da parte del concessionario, ma come non chiamare in causa chi ha regalato questo asset e non ha poi controllato il privato? I passati Governi hanno introdotto norme per cui controllato e controllore sono gli stessi. Il privato vuole il massimo guadagno con la minima spesa ed Autostrade è l’esempio più lampante: miliardi di fatturato e poche centinaia di milioni di investimenti per la manutenzione e la sicurezza. La gestione pubblica non funziona quando chi dirige non controlla o è corrotto. Lo slogan «privatizzare» è necessario alla scusa alla scusa per regalare ad amici e agli amici degli amici la cosa pubblica e ottenere favori e finanziamenti al partito e o direttamente dalle nostre tasche. Il crollo del ponte ha mostrato che decine e decine di ponti necessitano di interventi. Non si parla solo di ponti; le scuole, tutta la rete stradale e le gallerie

rivolta al Movimento è di aver perpetrato un condono. Che non sia così appare evidente se si legge il decreto-legge e si guarda il bene comune. A Ischia la norma è rivolta agli edifici che hanno subìto danni e che hanno pratiche di condono sospese. Le pratiche di cui si parla sono antecedenti al 2003. Chi ci ha preceduto e ha gestito la Regione Campania per anni e persino la maggior parte delle amministrazioni locali avrebbero dovuto chiudere queste pratiche e andare alla risistemazione degli edifici o, nel caso di mancata conformità, al loro abbattimento. Il mondo, però, è pieno di persone come Ponzio Pilato, che non si prendono le responsabilità che compete loro in quanto amministratori. Ischia è un ecosistema fragile e proprio per questo la ricostruzione necessita di un adeguamento sismico e del rispetto delle norme paesaggistiche, di sicurezza e sul dissesto idrogeologico, che sono previste nel Chi ha fatto una domanda allo Stato, anche oltre quindici anni fa, ha diritto a una risposta. Se ci sono domande sospese, queste impediscono di chiudere le pratiche aperte con il terremoto del 2017. Novembre 2018 di migliaia di edifici, come qualcuno ieri in Commissione ha vaneggiato. Si tratta di meno di mille edifici. Veniamo al terremoto del Centro Italia, dove sono state introdotte norme per una ricostruzione che, a oltre due anni di distanza, deve ancora decollare. A parte la nomina di un commissario, la struttura commissariale è stata semplificata e nella cabina di regia sono stati ammessi i sindaci. È stato previsto il compenso per amministratori di condomini e consorzi di proprietari. Significativo è l’anticipo del 50 per cento delle spese sostenute dai professionisti. Le ditte che effettuano indagini avevano smesso di farne perché, a fronte di una prestazione d’opera, non corrispondeva un rientro economico. Ci si chiede come sia possibile che siano stati spesi tanti miliardi e la ricostruzione sia ancora al palo. (Applausi soprattutto come siano stati spesi questi miliardi. Sono stati spesi in inutili sbancamenti e in opere di sistemazione e contenimento dei versanti per costruire casette di legno, che in questi giorni stanno ammuffendo e necessitano di trattamenti. Le famiglie terremotate stanno vivendo in ambienti insalubri e devono momentaneamente abbandonarli. Sono cifre stratosferiche, che arrivano fino a 6.500 euro al metro quadro. queste opere andranno demolite al termine dell’emergenza, con altre spese enormi per il ripristino dei luoghi. È stato puntellato di tutto e di più, inclusi edifici che avrebbero dovuto essere demoliti. 200.000 euro per puntellare. Ma che controlli hanno svolto il commissario e i subcommissari? È stato permesso che si potesse spendere senza alcuna gara e con compensi elevati per i progettisti senza ribassi d’asta. Ci sono stati i sindaci che, che, a fronte di una disponibilità di nuovo personale, hanno assunto amministrativi e avvocati e neppure un tecnico, come se tutta la partita si giocasse a livello burocratico. Ma quanti edifici sarebbero potuti essere ricostruiti con le centinaia di migliaia di euro utilizzati per i puntellamenti? Il condono è stato invocato anche per il Centro Italia. Tra le norme introdotte c’è quella che permette di regolarizzare le difformità fino al 20 per cento della cubatura quando non sono stati fatti interventi strutturali responsabili dei danni della struttura. Ci si dimentica che le Regioni, con l’introduzione del Piano casa, permettono di aumentare i volumi di un edificio fino al 20-30 per cento. Il PD in Commissione ha criticato i Piani casa, dimenticando che molte delle Regioni dove sono stati introdotti ed applicati sono gestite dal PD. In pratica, gli edifici con lievi difformità avrebbero dovu- to essere demoliti, ma poi, presentando la domanda in Regione, avrebbero potuto essere ricostruiti. Capisco che demolire e ricostruire fa circolare più denaro e quindi si ha più possibilità di dare incarichi e denaro pubblico agli amici. Ma dov’è il buon governo? La messa a norma avviene solo per gli edifici in cui viene garantita la stabilità a seguito di una perizia asseverata da parte di un tecnico. In Centro Italia, come Ischia, le porzioni di fabbricato che non erano a norma non ricevono denaro. Chiamare questo condono è pura ipocrisia.

Signor Presidente, ringrazio i relatori Ripamonti e Patuanelli perché hanno fatto un po’ di chiarezza - e altra ne faremo con gli interventi sulle bugie e sulle falsità, queste sì, che sono state sparse oltre i limiti del lecito dal PD nel Paese e anche oggi in Aula. Molto spesso ci rammarichiamo che i cittadini si fermino solo al titolo dei giornali o dei provvedimenti. Ebbene, almeno qui si dovrebbe fare qualcosa di più, senatore Ferrazzi, perché lamentarsi che su 46 articoli solo 11 parlino di Genova significa non aver letto che questo decreto-legge è anche il decreto Genova, oltre che il decreto sulla sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, sugli eventi sismici del 2016 e 2017 Bisognerebbe conoscere almeno il titolo, se non il contenuto del provvedimento: almeno questo, a chi siede in Parlamento, lo richiediamo, perché altrimenti significherebbe ingannare i cittadini. Queste emergenze hanno un filo che le unisce: il filo della responsabilità diretta o indiretta di coloro i quali ci hanno portati a questa situazione. Per mesi abbiamo sentito accusare

Risposte sui controlli e sugli interventi di un Paese le cui infrastrutture cadono letteralmente a pezzi, con la responsabilità di fornire una rete di impianti che eviti a monte l’emergenza, ad esempio, per i fanghi; risposte in termini di burocrazia. Venendo al merito, comincio - permettetemelo - dal terremoto del Centro Italia,

PD da un lato rivendicava i meriti dei commissari e dall’altro ci accusava di non fare abbastanza. Vorrei ricordare che in quella sede introducemmo delle prime risposte per le sanatorie pendenti e per le piccole difformità. Ebbene, nel corso di quella discussione, senatori Margiotta e Ferrazzi (potrei richiamare anche dopo la posizione del PD) non solo solo certe cose le avete dette, ma le avete scritte e le avete votate, perché l’emendamento 1.75 a firma Verducci, Ginetti, Grimani, che tutti i senatori del PD presenti votarono, recitava (ne leggo solo alcuni passaggi): «In presenza di edifici danneggiati da eventi sismici, per i quali in conseguenza di istanza di condono ai sensi delle leggi n. 47 e n. 326 del 2003,» - guarda caso le stesse citate dal senatore Ferrazzi - «il Comune non ha provveduto al rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, la certificazione di idoneità statica o sismica, ove richiesta ai fini della concessione medesima, può essere sostituita dall’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione preposta al vincolo sismico, in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dell’edificio danneggiato,

in assenza del permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata (…) o in difformità da essa, il proprietario dell’immobile, pur se diverso dal responsabile dell’abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo (…)», eccetera eccetera eccetera. senatore Ferrazzi, voi non è che cambiate idea solo da quando siete in maggioranza a quando siete in minoranza, ma cambiate idea anche da quando siete in minoranza a quando siete in minoranza. Vorrei anche ricordare - l’ha già fatto il collega Coltorti - che i Presidenti delle Regioni Umbria e Marche, ad esempio, chiedevano quello che noi oggi, come avevamo promesso, abbiamo completato, con l’individuazione del 20 per cento di massima difformità e non prevedendo contributi per quanto riguarda gli

regionale e nazionale, ha governato e non ha fatto o non ha fatto in modo che altri facessero. Ometto l’elenco del colore politico dei sindaci, dei Presidenti di Regione e dei Governi, per esigenze di tempo. esigenze di tempo. Chiudere un condono significa dare risposte, abbattere quello che c’è da abbattere e sanare quello che c’è da sanare. E lo facciamo in maniera ancora più restrittiva, perché sul piano dei soggetti non tutti potranno richiederlo (chi ha avuto condanne per associazione mafiosa non potrà farlo) e non tutto potrà essere sanato

onorevoli colleghi, prima di ogni cosa è doveroso - credo per tutti noi - esprimere sentimenti di vicinanza e solidarietà ai cittadini di Genova e a quanti hanno perso, in quel tragico crollo, familiari e amici. Siamo tutti accanto a voi e sono certo che la città, sostenuta da un popolo fiero, coraggioso e determinato, troverà la forza di ripartire. A noi sta il dovere morale e politico di non lasciarvi soli e di accompagnarvi nel modo migliore in questo difficile cammino. Il decreto-legge quest’Assemblea si appresta ad approvare contiene una serie di misure significative e molto importanti, che rispondono a esigenze di diversi territori, risposte a situazioni molto complesse e ad eventi imprevedibili, così come a situazioni per le quali, Grazie! Il testo interviene concretamente per far fronte a situazioni emergenziali. Anche in questa sede va quindi dato atto all’Esecutivo del lavoro svolto con determinazione e velocità. Fare presto e fare bene è stato il paradigma che ha guidato l’azione del Governo negli ultimi mesi, in questa come in tante altre circostanze. (Com_menti della senatrice Pinotti). Affermare il contrario, come fatto in queste_ settimane da alcuni colleghi dell’opposizione, sarebbe da ascrivere a mera propaganda, finalizzata poi a non si sa bene quale illusorio tornaconto. Io capisco che si tratti di percezione, sensibilità umana, sensibilità politica, di contatto con la realtà. Qualcuno, forse, questo contatto lo ha perso: forse, dal Gruppo M5S). Tuttavia consiglio di non ricercare questo contatto attaccando il lavoro di chi si è adoperato e si adopera, come nel caso di questo decreto-legge, per sopperire ad anni ed anni di incuria e di totale disinteresse. Anni in cui si è preferito voltarsi dall’altra parte e far finta di non vedere per scaricare su altri le responsabilità di mancanze ed inadeguatezze di una classe politica malata, indifferente, sorda e arroccata su posizioni indifendibili. Oggi qui finalmente stiamo dando degli strumenti, fondi ai territori, alle imprese e ai lavoratori. Dite che siamo contrari alle opere e alle infrastrutture, che blocchiamo il Paese, questo è il vostro mantra quotidiano. (Proteste

Con una tabella di marcia definitiva e con obiettivi a medio e lungo termine, fronteggiando le emergenze come in questo caso. In pratica, stiamo evitando di fare ciò che avete fatto voi.

Un accenno al ben noto caso della messa in sicurezza della A24 e la A25, visto che sono abruzzese, voglio farlo. Dopo dieci anni di nulla assoluto, sentire le accuse mosse alla maggioranza e al Governo ha veramente del ridicolo. A quanti nel PD abruzzese, e anche nazionale, hanno cercato con ogni mezzo a loro disposizione di fornire una visione distorta dei fatti, io rispondo con le misure concrete contenute in questo provvedimento che arriva, lo ripeto, dopo dieci lunghissimi anni di nulla assoluto. I frutti di questo nulla li raccoglierete, così come li avete raccolti il 4 marzo, anche alle regionali di febbraio 2019. (Commenti del senatore Fara_one)._ Tornando alle misure contenute nel provvedimento, desidero esprimere particolare soddisfazione non le motivazioni già elencate e richiamate ma anche per alcune particolari disposizioni che vanno, a mio modesto avviso, nella giusta direzione. Mi riferisco al sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza, alla istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, delle infrastrutture stradali e autostradali e all’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche. Non c’era niente. Gli obiettivi che abbiamo intenzione di raggiungere con queste misure sono diversi: garantire elevati standard di sicurezza e avere contezza e immediati riscontri su dati tecnici, stato e grado di efficienza delle opere, sull’attività di manutenzione ordinaria e sullo stato dei lavori. Insomma, sul tavolo, finalmente, ci sono strumenti e soluzioni per gestire l’emergenza e per voltare decisamente pagina rispetto al passato. Un grazie va rivolto un grazie ai cittadini parlamentari del MoVimento 5 Stelle e un grazie ai colleghi della Lega per aver lavorato con l’obiettivo di assicurare una migliore e sempre più efficiente gestione del territorio, delle infrastrutture e delle risorse. Colleghi, visto che ho ancora un po’ di tempo, mi rivolgo a chi ieri sera ha dato appiglio all’opposizione per intervenire su un tema che non c’è. Li facciamo parlare di un condono che non c’è.

non c’è risposta, come c’è stato negli ultimi trent’anni perché i sindaci che avete non avevano il coraggio di prendere una decisione, ci sarà il silenzio-rigetto.

Dunque, colleghi della maggioranza, del MoVimento 5 Stelle e della Lega, stiamo andando alla grande: avanti così. È iscritto a parlare il senatore Nastri. Ne ha facoltà.

Vorremmo ricordare al ministro Toninelli, ancora una volta assente da quest’Aula che, se questo decreto-legge fosse stato scritto bene, sarebbe già in vigore e, se oggi è così importante, è perché, così facendo, diamo almeno delle regole certe, discipliniamo, evitando al commissario, al sindaco Bucci,

alla fine, invece, abbiamo un coacervo di norme astruse, oltre che eterogenee, e per nulla in sintonia con l’originaria finalità. Il decreto Genova ambiva a essere una legge speciale, mentre quello che stiamo per votare non è il decreto per Genova, né una legge speciale per Genova, come già È un decreto per così dire «macedonia», nel quale hanno trovato spazio tante altre emergenze, terremoti vicini e lontani, tragedie recenti

complete. Sono mancati - come detto - il coraggio e una visione, due categorie che distinguono la classe politica della bassa manovalanza da quella che invece ha una visione più ampia rispetto a quella che state dimostrando oggi. il tempo che abbiamo avuto di disposizione per l’esame dei 46 articoli è stato molto stretto, considerando che il decreto-legge deve essere convertito entro la fine di questo mese. Il Gruppo Fratelli d’Italia, sia alla Camera che al Senato, ha avuto sin dall’inizio

Mancava, soprattutto nella prima parte del decreto-legge, la componente più importante, quella dedicata ad affrontare l’emergenza e la situazione di Genova, sia per gli sfollati che per l’abbattimento e la ricostruzione del ponte. Certo, non si può non evidenziare in questa sede come il testo contenga norme che nulla c’entrano con Genova,

a vigilare. Non ci fermeremo nel denunciare norme come quelle previste da questo decreto-legge, che introducono e bisogna dirlo - una sanatoria applicabile in assenza di qualsiasi richiesta di autorizzazione passata, con un limite di tolleranza

una nuova stagione di controllo, vigilanza, manutenzione e ricucitura di un Paese ferito, che vede i suoi ponti crollare e le sue infrastrutture tremare, avremmo dovuto

un’intera economia, quella portuale, che riguarda lo scalo marittimo forse più importante in Italia, i cui armatori, non solo genovesi, stanno già dirottando le loro merci verso Marsiglia e Barcellona. Genova e l’Italia forse meritavano una risposta più veloce, certa e rassicurante. I nostri emendamenti, sia alla Camera che al Senato, andavano proprio in questa direzione,

inizialmente per gli sfollati e le persone che hanno perso la casa, che si sono giustamente indignate per una tale disattenzione e mancanza di risposta da parte del Governo. A un certo punto abbiamo fatto i conti

In tutto questo abbiamo cercato di dare il nostro contributo, anche se i nostri emendamenti sono stati purtroppo bocciati completamente.

fatti che hanno avuto la loro genesi in periodi lontani o mediamente lontani, come ad esempio lo sciame sismico, iniziato nel 2016, che ha duramente colpito quattro Regioni del Centro Italia e che - ricordo a tutti - è ancora in corso. Non è solo l’attualità dell’evento, però, che giustifica appieno la presenza dell’urgenza, ma anche - tutti ricordano sempre

e l’impossibilità di vedere una prospettiva e un proprio futuro in una situazione che lo Stato aveva il dovere di risolvere, ma che purtroppo ha pesantemente peggiorato.

soluzioni che avrebbero dovuto essere adeguate a ospitare le persone per il periodo necessario alla ricostruzione e che, dopo pochi mesi dalla loro realizzazione, già stanno marcendo: stanno marcendo i soffitti e i pavimenti. si stanno dimostrando del tutto inadeguate a quello che era il loro scopo. E, se questa non è urgenza, allora vorrei proprio capire che cosa sia una urgenza per i colleghi del Partito Democratico, che sono arrivati anche a insinuare

Dov’è l’etica nel non dare risposte a persone che chiedevano solo quello? Dov’è l’etica nel bocciare e bloccare una ricostruzione che sarà, probabilmente, la più importante fatta in Italia? E dov’è l’etica nel non consentire, a chi è pienamente titolato a ricostruire, di farlo? Se tutti puntano il dito nei confronti delle poche irregolarità presenti nel Centro Italia, nessuno ricorda che quelle poche irregolarità bloccano anche chi quelle irregolarità le subisce. La ricostruzione, infatti, verrà fatta per aggregati: più persone che per esigenze tecniche dovranno ricostruire insieme e che insieme si trovano bloccate, spesso per una problematica che non incide in alcun modo sulla sostanza e sulla solidità dell’edificio ma che, per problemi amministrativi, blocca la ricostruzione. È questo quello che stiamo facendo noi: non un nuovo condono, come colpevolmente e irresponsabilmente alcuni colleghi del Partito ma semplicemente stiamo dando risposte. È vero, infatti, che il condono non è un diritto, ma lo è avere le risposte; ed è un diritto talmente acclarato che si è arrivati anche

che la risposta è un diritto e ci stiamo prendendo la responsabilità di dare risposte, come previsto all’articolo 25, che voglio leggere perché - come ha già detto prima un collega - la superficialità e la banalità di certi interventi si fermano

Si ipotizzava poi la possibilità di andare a premiare chi era in una situazione di irregolarità.

Quella che sarà ricordata come la peggiore ricostruzione della storia, ancora al palo dopo due anni, noi stiamo cercando faticosamente di far ripartire farla ripartire con il buonsenso. Siamo stati accusati di aver leso le prerogative delle Regioni perché abbiamo previsto espressamente che il commissario possa solo comunicare alle Regioni le proprie ordinanze. Sono sessantanove le ordinanze da rimodulare. vorrei proprio vedere come chi ha adottato quelle ordinanze, cioè le Regioni - come è stato fatto - possa avere un ruolo attivo

a imprese e lavoratori; sostiene il trasporto pubblico locale, la logistica del porto, la sua ripresa e il suo sviluppo. Inoltre, promuove eccezionali misure di sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, istituendo un’agenzia per la sicurezza, un archivio informatico per le opere pubbliche e un sistema di monitoraggio dinamico delle infrastrutture. Per la prima volta in Italia l’emergenza si trasforma in prevenzione. È la rivoluzione culturale di questo Governo con tre prodigiose S: sostegno, sviluppo e sicurezza. Nelle altre emergenze si superano inefficienze e ritardi accumulati in un decennio da ben cinque Governi negli ultimi cinque terremoti distruttivi italiani. L’articolo 25 non è un condono. Dopo biasimevoli condoni edilizi e pessime ge- stioni dell’abusivismo - ancora in atto - non sono tollerabili comportamenti politicamente dissociati e palesemente strumentali. Non è un condono. Per il primato della verità, è definizione delle procedure di condono, ferme da decenni, al fine di accedere ai contributi per la ricostruzione, nell’ambito di programmi di riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico. Negare all’infinito una risposta declassa i richiedenti a figli di un Dio minore. In Commissione è stato narrato come mezzo di distruzione di massa, perché si condonerebbero decine di migliaia di case abusive mal costruite. È esattamente il contrario. Definire le poche pratiche di condono contemplate, per consentire a chi ne ha i requisiti, e nel rispetto dei vincoli paesaggistici, di accedere ai contributi, significa rendere più sicuro il patrimonio edilizio. Da geofisico, vi dico che i frequenti terremoti ischitani, deboli nella magnitudo ma molto forti nello scuotimento, non suonano il campanello quando arrivano. E, se trovano case vulnerabili, a causa di lentezze burocratiche, le abbatteranno, persone comprese. L’articolo 25 sancisce un diritto e può salvare la vita. Passo all’articolo 41 che reca disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione. In un assordante silenzio politico, si sono tollerate pratiche agricole aggressive e velenose. Dove erano gli attuali improvvisati censori negli ultimi ventisei anni, alle Bahamas? decreto legislativo n. 99 del 1992 che consente e regola lo spandimento dei fanghi su suoli agricoli. In quel decreto gli idrocarburi pesanti C10-C40, così come molte altre sostanze tossiche e cancerogene, non sono tabellati. La Regione Lombardia fissò per gli idrocarburi pesanti un limite di 10 grammi per chilogrammo di sostanza secca. Ci fu un ricorso e, a luglio scorso, il TAR stabilì che per C10-C40

Pur comprendendo la ratio della sentenza, il limite di cui sopra ri- guarda il sistema suolo, composto da terra più inquinante. Il limite del TAR, applicato al solo fango, avrebbe difatti impedito un suo spandimento, con gravi problemi di stoccaggio temporaneo e necessità di trattamento, messa in discarica o incenerimento immediato. L’articolo 41 rimedia a tale grave emergenza. Per gli idrocarburi pesanti, considerando che non tutti sono cancerogeni e sono naturalmente presenti nella sostanza organica, il limite di 50 milligrammi è di fatto attualmente improponibile. Da esperto di monitoraggi geofisici per l’agricoltura di precisione, vi dico che gli idrocarburi si formano anche naturalmente nei suoli agrari e forestali. La semplice caduta delle foglie in un bosco può causare concentrazioni di idrocarburi ben superiori al limite di 50 milligrammi per chilogrammo, come la letteratura internazionale sancisce.

per chilogrammo di tal quale. Ciò significa che nel sistema suolo interessato dallo spandimento, il fango peserà al massimo per una decina di milligrammi per chilogrammo di sostanza secca, al netto di assorbimenti vari,

toluene, selenio, berillio, arsenico, cromo, eccetera. Verranno finalmente monitorati e non permessi. Quindi, il decreto-legge garantisce maggior sicurezza sulla provenienza e sulla qualità dei fanghi: facciamo un notevole passo in avanti. Siccome in Commissione si è poi narrato di spandimenti scriteriati di fanghi su colture in atto, quasi che fossero sparsi - non so - su insalata e pomodori, tengo a dire che, in tal caso, essi sono vietati legislativo, così come in colture orticole e frutticole nei dieci mesi antecedenti il raccolto. Comunque, l’incipit dell’articolo 41 è «Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore,» eccetera. La normativa come ha detto bene il relatore e come più volte ha ribadito il ministro Costa - sarà rivista. Non faremo gli struzzi come chi ci ha preceduto. Anche nel caso dei fanghi, siamo dalla parte dell’ambiente, di un’agricoltura sana e della vita, ma decisamente contro le falsità e le strumentalizzazioni.

tutti temono - o altro non importa. Parliamo di zone che versano in una situazione di emergenza, dove la ricostruzione non va avanti perché le case non hanno i titoli abitativi.

Signor Presidente, onorevoli senatori, ancora oggi, mentre parliamo in questa sede, migliaia di nostri concittadini sono in enormi difficoltà, fuori dalle proprie case e con enormi incertezze sul proprio futuro, e questo dopo oltre due anni dall’inizio degli eventi sismici dell’agosto del 2016. Già il fatto che, dopo oltre due anni, stiamo ancora parlando di emergenza, oltre che una distorsione della lingua italiana, è un segno inequivocabile e incontestabile dell’ennesimo fallimento della classe politica che ci ha preceduto. Il fatto che delle critiche al provvedimento in esame arrivino proprio da lì, da chi ha gestito finora la ricostruzione, con risultati purtroppo pressoché inesistenti, e dopo aver proposto provvedimenti ben più permissivi del nostro, è invece il segno inequivocabile che questa classe politica ha definitivamente perso di vista il bene dei cittadini, oltre che la realtà. Il nostro provvedimento nasce invece proprio dall’ascolto dei problemi reali riportati da cittadini, ordini professionali, esperti di tutela del territorio e amministratori locali. E non è un caso che sia stato accolto molto favorevolmente, come una liberazione, addirittura anche da governatori di Regioni Già solo questo dovrebbe mettere fine a ogni polemica. Invece, dobbiamo assistere a un ultimo tentativo di ritardare ancora quella ricostruzione che permetterebbe, finalmente, a decine di migliaia di nostri concittadini di ricominciare una vita normale e alle casse dello Stato di risparmiare sui costi delle sistemazioni autonome, stimolando al tempo stesso l’economia delle zone colpite attraverso il traino dei settori coinvolti, a partire ovviamente dall’edilizia. Negli ultimi giorni - e anche oggi - si è fatto un gran parlare della questione dei cosiddetti condoni, difformità o abusi presenti nei fabbricati colpiti dal sisma.

Pertanto, dobbiamo tenere ben presente che stiamo parlando di cittadini italiani che hanno presentato un’istanza legittima, secondo leggi approvate in quest’Aula e sicuramente non da questa maggioranza.

danni non solo puramente economici ai cittadini. Quando, nella situazione di emergenza attuale, in attesa di una ricostruzione bloccata dalla burocrazia, in molti non possono rientrare nella propria abitazione, la vita risulta stravolta.

Non posso che dichiararmi soddisfatto per il buon senso che da sempre contraddistingue l’azione di questo Governo, che ha come sola e unica bussola l’interesse dei cittadini. Aggiungo qualche annotazione da tecnico con esperienza nella pubblica amministrazione: sono consapevole che il patrimonio edilizio del nostro Paese, e in particolare quello del Centro Italia colpito dal sisma, è composto da un tessuto immobiliare di enorme valore storico e artistico, oltre che fragile. So bene che l’epoca di costruzione di molti edifici non è riconducibile alle norme edilizie e urbanistiche recenti,

con poi il sistema di vincoli introdotto dalla legge n. 431 del 1985, il Testo unico n. 380 del 2001 e la legge n. 42 del 2004; una ragnatela di normative che, per ragioni varie, non tutti i Comuni hanno attuato e recepito con la stessa tempestività. So bene quindi, per averlo vissuto dall’interno, che la situazione della conformità amministrativa del patrimonio immobiliare è estremamente complessa, non tanto per le difficoltà di attuazione della normativa, ma ancor di più per decenni di mancato controllo del territorio, per provvedimenti non adottati da una burocrazia farraginosa, oltre che per quei privati che di questa situazione ambigua hanno anche cercato di approfittare. Ma è ora di ripartire. Con l’articolo 25 sblocchiamo la ricostruzione delle aree colpite nel 2017 dal sisma di Ischia: acceleriamo le procedure in modo che entro sei mesi, dopo trent’anni di attesa, chi aveva fatto in passato richiesta di condono riceva un sì o un no. I proprietari delle mille case danneggiate dal sisma aspettano da trent’anni di sapere che destino avrà la loro abitazione e ora se hanno diritto ai fondi per la ricostruzione. Se la richiesta viene respinta i proprietari, non riceveranno neanche un euro per la ricostruzione. Se la richiesta è accolta, riceveranno i contributi, ma non per le nuove volumetrie costruite abusivamente. Nessun contributo invece va a chi è condannato per mafia e riciclaggio di denaro sporco. In ogni caso, non ci sarà alcun nuovo condono: un rischio paventato solo da una comunicazione scorretta, centrata su un falso scontro ideologico politico e purtroppo lontana dalla ricerca di soluzioni concrete per i cittadini. Dopo due anni di blocco totale della ricostruzione, siamo in grado di dare una buona notizia alle persone che nel Centro Italia fanno i conti ogni giorno con i danni del terremoto: nel cosiddetto decreto emergenze si sblocca il freno rappresentato dalla presenza di centinaia di piccole e limitate difformità edilizie, con una norma capace di far ripartire i cantieri e sbloccare la possibilità di utilizzare i fondi stanziati per la ricostruzione. Chi chiede il contributo dimostrando che la propria abitazione ha subìto danni potrà anche chiedere la regolarizzazione per le piccole modifiche realizzate decenni fa, molto spesso ricevute in eredità insieme alle case di nonni e genitori. Saranno regolarizzati anche gli aumenti di volumetria che oggi sono ammessi per legge, perché rientrano nelle norme regionali sul Piano casa, fermo restando che su questa volumetria aggiuntiva il contributo per la ricostruzione non verrà riconosciuto. francamente la logica di una polemica - a mio giudizio puramente strumentale - per cui una norma che porta vantaggi volumetrici oggi è cosa buona e giusta - mi riferisco ancora al Piano casa - mentre, se la stessa viene applicata per far rinascere un territorio in difficoltà, è da osteggiare. Questo, signor Presidente, Tanti Comuni del cratere sono borghi storici che noi amiamo profondamente e conosciamo: nelle case di quei centri si sono stratificate, nei secoli, piccole difformità che hanno reso impossibile riconoscere ai proprietari il contributo per la ricostruzione, secondo norme evidentemente scritte senza conoscere le realtà a cui andavano applicate. Parliamo di finestre murate, di porte allargate di qualche centimetro: veramente inezie. Finalmente abbiamo eliminato questo ostacolo, pur conservando la garanzia dei massimi standard di sicurezza e tutela dell’ambiente e del paesaggio: ogni intervento di ristrutturazione e di ricostruzione sarà fatto verificando la sicurezza statica e antisismica degli edifici e - ricordiamolo - per le strutture totalmente abusive non ci sarà alcuna sanatoria. non diamo soldi pubblici ai furbi e tuteliamo invece i cittadini vittime di un ingranaggio inceppato. Siamo orgogliosi di poter dire che, grazie al nostro lavoro, la ricostruzione finalmente parte: uno dei passi necessari per trasformare l’Italia da Paese delle emergenze a Paese organizzato su modelli di qualità che tutelano tutti i cittadini.

Signor Presidente, onorevoli colle- ghi, il 7 ottobre 1970 Genova fu sommersa da un’alluvione di rara potenza, con morti, feriti e sfollati. Nella zona di Sant’Agata crollò il ponte medievale sul Bisagno. Tant’è che ancora oggi ne possiamo vedere in parte le rovine come un monito alla prevenzione contro il dissesto idrogeologico. Un monito rimasto inascoltato. Infatti, nel 2011 e nel 2014 Genova ha nuovamente pianto le sue vittime.

Ma il 14 agosto 2018 è capitato qualcosa di molto diverso dalle tragedie che Genova tristemente ha imparato a conoscere. Qui la natura non c’entra nulla, neanche minimamente, nel crollo del viadotto Morandi. Ogni responsabilità è in capo all’uomo e da questo punto di vista il crollo del ponte assume un’aura sinistra. Qualcuno non ha vigilato; qualcuno è venuto meno ai suoi doveri; qualcuno dovrà pagare. PSd’Az). In più occasioni abbiamo elogiato l’incredibile reazione della macchina dei soccorsi, della Protezione civile, dei Vigili del fuoco, del Sistema sanitario e dei semplici cittadini, che durante e all’indomani dei disastri si trasformano puntualmente in anonimi eroi a cui non può non rivolgersi il nostro riconoscimento. Ogni ulteriore parola a questo riguardo è superflua, perché, come ha dichiarato il ministro Salvini parlando dei Vigili del fuoco, le pacche sulle spalle non bastano più. Il momento dei fatti concreti è finalmente arrivato e il decreto Genova oggi in discussione è un provvedimento la cui concretezza traccia un’enorme linea di demarcazione e di discontinuità con gli analoghi provvedimenti che i Governi passati hanno varato all’indomani delle calamità naturali o dei disastri artificiali. La discontinuità è il tratto saliente del decreto Genova. Discontinuità che, improvvisa e inaspettata forse agli occhi degli osservatori internazionali e nazionali, è sorta fin dalle prime ore del disastro. Infatti, si è visto subito all’opera un nuovo modo di fare politica amministrativa, di gestire l’emergenza e di affrontare le ricadute psicologiche sulla popolazione. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, nominato commissario straordinario all’emergenza, insieme al sindaco Bucci, non a caso nominato successivamente commissario straordinario per la ricostruzione, sono stati presenti sul territorio fin dal primo momento, affiancando l’operato del Governo nazionale, che in maniera costante costante e puntuale non ha mai abbandonato Genova, sia attraverso l’operato quotidiano del vice ministro genovese Edoardo Rixi, che non ha mai lasciato per un secondo la sua terra e la sua gente e che per questo ringrazio. sia attraverso la presenza del presidente del Consiglio Conte, dei vice premier Salvini e Di Maio e del ministro Toninelli. Discontinuità c’è stata nella volontà di additare subito i colpevoli, senza cadere nel circolo vizioso tipico della vecchia politica di fare dichiarazioni di principio che non portano a niente. Discontinuità c’è stata nella gestione degli sfollati che, a differenza dei nostri connazionali colpiti dal terremoto del Centro Italia, non subiranno l’umiliazione e il disagio di passare un inverno al freddo nelle tendopoli. E infatti, nessun caso come quello di nonna Peppina Peppina si è verificato a Genova. Discontinuità c’è stata nell’immediata opera di intervento sugli integrati sistemi logistico, produttivo, industriale e commerciale danneggiati dal crollo del viadotto. Discontinuità c’è stata, infine, nel rapporto emotivo e simpatetico tra le istituzioni e il popolo, qualcosa cui l’Italia non era più abituata da molto tempo. Novembre 2018 della discontinuità è ora il momento di ripartire e il decreto Genova offre gli strumenti e le risorse necessarie a farlo. Un miliardo di euro arriverà sul territorio. Niente è lasciato al caso. Vorrei trattare brevemente alcuni punti su cui ritengo sia bene porre l’accento perché rappresentativi dello spirito fondante del decreto in discussione. L’attenzione per gli sfollati è stata confermata in tutta la sua portata. Il valore dei loro immobili sarà calcolato attraverso lo strumento del Programma regionale di intervento strategico, con un ulteriore incremento del valore risultante, perché è giusto che anche l’aspetto emotivo della perdita sia tenuto in considerazione. infatti, lasciano la loro storia personale, i loro ricordi e le loro paure all’interno di quelle mura. Il perimetro amministrativo nel quale si iscrivono i poteri del commissario è stato delineato per garantire la razionalità e l’efficienza delle decisioni. Grazie all’istituzione di una zona franca che va nella direzione auspicata da più parti nei giorni immediatamente successivi al crollo del viadotto, le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all’interno di esso o che hanno subìto, a causa dell’evento, una riduzione del fatturato possono richiedere alcune agevolazioni in alternativa agli altri benefici previsti. In ultimo, il decreto per Genova lancia un messaggio chiaro al Paese: la tragedia del Morandi non può non avere ricadute sensibili sull’attenzione che le istituzioni hanno nei confronti della manutenzione Un crollo come quello del Morandi non deve più ripetersi. Sarà realizzato un sistema sperimentale di monitoraggio dinamico, a cui sovrintenderà il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

In occasione dei funerali di Stato i rappresentanti del Governo sono stati applauditi, mentre qualcun altro è stato fischiato. Quegli applausi sono stati una dimostrazione spontanea e calorosa di fiducia e rappresentano una responsabilità enorme, perché questa maggioranza è chiamata a non deludere chi ha mostrato di credere in lei. Il decreto Genova va in questa direzione, è un passo in avanti verso una ricostruzione che non potrà cancellare il dolore, ma potrà farci diventare più forti di prima. Oggi non Oggi non vi sono alibi né scuse per non votare questo decreto: è quello che dobbiamo a Genova e che dobbiamo a tutta l’Italia. (Applausi

il decreto-legge a cui stiamo dando conversione contiene misure concrete per la città di Genova e per i genovesi,

e si ristabilisce quel giusto equilibrio che spetta all’interesse pubblico. Infatti, tra gli interventi previsti ce n’è uno che prevede l’acquisizione del parere da parte dell’Autorità di regolazione dei trasporti nei casi di aggiornamento e revisione delle concessioni autostradali in essere, in modo da poter riequilibrare quelle condizioni contrattuali che oggi risultano essere eccessivamente favorevoli agli interessi del privato e a discapito dell’interesse pubblico. Oggi lo Stato è tornato a fare lo Stato e con questo provvedimento ne dà piena dimostrazione. Mi sento in dovere di ringraziare il ministro Toninelli, anche a nome di tutti i cittadini abruzzesi per il particolare interesse che ha riservato alle gravi condizioni di sicurezza dei viadotti delle autostrade A24 e A25. (Applausi dal Gruppo M5S). Autostrade definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2003 di interesse strategico, per le finalità di protezione civile in caso di eventi sismici, ma che, ciò nonostante, risultano interessate da un grave stato di ammaloramento nei piloni che sorreggono le stesse strutture. Il Ministro si è recato di persona a constatare la fragilità di quei viadotti, dove cadono pezzi di calcestruzzo e i tondini dell’armatura, arrugginiti e completamente scoperti dalla malta cementizia, gli si sono spezzati tra le mani come fossero biscotti. Nonostante la campagna strumentale portata avanti da alcuni politici del territorio (quelli bravi ed esperti, quelli che hanno lasciato marcire quell’autostrada) il Ministro ha trovato il modo di dotare l’urgenza di uno stanziamento di 196 milioni di euro per dare avvio a quella manutenzione che mai - e dico «mai» - era stata fatta. E ancora: è prevista l’assunzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di 110 tecnici, dedicati ai sopralluoghi ed al controllo di tutte le infrastrutture, in modo che mai più possa verificarsi una tragedia come quella dello scorso 14 agosto, avvenuta a Genova. All’interno del decreto emergenze viene prevista l’istituzione dell’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, attraverso il quale sarà possibile identificare univocamente ciascuna struttura presente sul territorio nazionale, grazie anche alla possibilità di consultazione dello stesso archivio, in formato open data. Avremo insomma nuovi strumenti di prevenzione, di cui tutti i cittadini potranno godere in termini di sicurezza. Inoltre, inizierà un’importante fase di monitoraggio sperimentale per le opere ritenute prioritarie, mediante un sistema dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità. Si tratta di un controllo strumentale costante delle infrastrutture stesse, che si avvarrà dell’ausilio delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali. Questo strumento contribuirà inoltre a rendere più agevole il processo di programmazione, finanziamento e priorità degli interventi da eseguire sulle opere. Per questi e per tutti gli altri interventi previsti nel decreto-legge n. 109 oggi in conversione non finiremo mai di ringraziare questo Governo.

non tornerò sulle cose già condivise che motivano l’opposizione precisa e pervicace a questo doppio condono, che offende non soltanto i cittadini in regola, ma in particolare, in questo caso, la città di Genova. Non ho molto tempo a disposizione, quindi toccherò due problemi e due questioni sui quali non si è, secondo la mia opinione, approfondito a sufficienza. Il decreto-legge per Genova era l’occasione per costruire uno scenario che mettesse o confermasse la città di Genova al centro di un quadrante che la caduta del ponte aveva irrimediabilmente messo in difficoltà. Il decreto-legge arriva con colpevolissimo ritardo (novanta giorni dopo i fatti drammatici che hanno colpito la città); ma soprattutto, in questi novanta giorni, si è costruito attorno alla città di Genova una sorta di deserto, che rischia di mettere in crisi in maniera decisa e temporalmente terribilmente efficace il futuro di un quadrante indispensabile allo sviluppo dell’Italia, non solo allo sviluppo di una Regione. Da una parte è stata messa in discussione la realizzazione del terzo valico, c’è la conferma del «no» alla Gronda e soprattutto, a corredo di quel quadrante geostrategico dal punto di vista sociale e dal punto di vista economico, c’è la conferma del «no» alla Torino-Lione. La somma di tutti questi fattori non incide soltanto sul porto di Genova, ma mette il porto di Genova, con il quadrante di riferimento (cioè soprattutto il suo entroterra), di creare un guasto irreversibile per la crescita di tutto il Nord italiano e quindi di larga parte di questo straordinario Paese. Ha ragione il presidente Coltorti, quando fa appello alle carenze dei Governi precedenti. Il presidente Coltorti si è invece dimenticato di specificare quali siano i Governi precedenti. Glielo ricordo molto volentieri: tra il 2008 e il 2013 (non governava il centrosinistra) gli investimenti sono decresciuti del 33 per cento (sono dati dell’ANCE, non sono dati di parte). La Lega - questo è un dato oggettivo, basta rileggersi le carte parlamentari - approva nel 2008 il protocollo con Autostrade, che conferma quella tipologia di concessioni. L’ultimo dato, invece, lo traggo dal CRESME: tra il 2013 e il 2018 i Governi uscenti hanno lasciato sul tavolo 149 miliardi (non 150) di investimenti legati a opere pubbliche, sia per la manutenzione, sia per le grandi infrastrutture. sono numeri, presidente Coltorti, che la prego di smentire con le carte alla mano; le mie carte sono qui e gliele farò avere molto volentieri, quando me ne farà richiesta. L’ultima questione riguarda un punto centrale del decreto Genova. Tutto viene derogato: si deroga nella gestione dei rifiuti, si deroga in termini di sicurezza del lavoro, si deroga in termini di appalti.

prevedeva la soluzione più puntuale e trasparente. Anziché mettere in discussione un apparato straordinario di leggi dello Stato,

Come gestirete le altre emergenze, in testa l’emergenza Veneto o l’emergenza che si è aperta con le alluvioni recenti in altre Regioni? Deroghiamo diversamente rispetto alle norme che avevamo circa la gestione e il governo della questione Genova? Oppure quello diventa il criterio da applicare anche alla gestione di altre emergenze? È ignoto. Il rischio, di fronte all’ignoto, è che cancelliate alcune norme e che altre rischino di non avere pienamente diritto di cittadinanza, sommando quindi ritardi colpevoli a ritardi ancora più colpevoli.

Presidente, nel breve tempo che ho a disposizione vorrei concentrarmi su due articoli, cioè il 25 e il 41, che non mi aspettavo, ovviamente, di trovare in un decreto-legge che doveva essere dedicato all’emergenza di Genova. Purtroppo, come spesso mi accade, il mio discorso toccherà in parte anche cose dette da altri colleghi perché, onestamente, non c’era bisogno di dirle: si potevano difendere gli articoli 25 e 41 senza ricorrere a queste affermazioni. premessa, per quanto riguarda l’articolo 25, possiamo anche non chiamarlo condono, però la domanda alla quale rispondere è la seguente: a legislazione vigente, quante abitazioni sull’isola di Ischia sono sanabili attualmente? La risposta è zero. Con questo articolo, quante abitazioni saranno sanabili? Più di zero. L’aritmetica di base ci dice che qualunque numero maggiore di zero è un numero positivo e quindi ci saranno delle case sanate, questo è molto semplice. Quante non lo so. secondo luogo, giustamente è stato detto che il condono non è un diritto, perché non lo è, ma il cittadino ha il diritto di avere una risposta al processo amministrativo che lo riguarda. Ma quale cittadino? Perché, limitandosi solamente alle abitazioni che riguardano i tre Comuni del comprensorio di Ischia che hanno avuto danni, restano escluse circa 844.000 istanze di condono su tutto il territorio nazionale. Queste persone hanno, anche loro, pratiche in corso alle quali non si dà risposta, quindi creiamo una dissimetria tra chi avrà una risposta e chi no. Ovviamente, possiamo estendere a tutti i cittadini che aspettano una risposta in trenta, sessanta, giorni e non ce l’hanno. Queste persone, evidentemente, non hanno un Santo a cui votarsi e quindi non avranno risposta. Inoltre, è stato detto che non ci sarà un contributo per la ricostruzione per coloro che hanno fatto incrementi di volumetria. Ci mancherebbe altro, dico io.

edifici in tutto o in parte costruiti in un’economia a nero, perché nessuna azienda fattura i lavori per una casa che è costruita abusivamente, senza i necessari requisiti di staticità, perché non sono state espletate tutte le procedure tecniche. Sono case costruite al risparmio,

e sarebbe anche il caso di farlo. È stato anche detto che ci sarà il silenzio-rigetto, ma non c’è scritto, nell’articolo 25 non compare. In compenso, esiste l’emendamento 25.25 (testo 2) che chiede esplicitamente il silenzio-rigetto ed è stato respinto in Commissione.

che il decreto legislativo n. 99 del 1992 non disciplina i livelli limite di dispersione di determinate sostanze, ma non è vero.

Ho anche sentito dire che adesso saremo tutti contenti, perché verranno dispersi sui campi dei fanghi con livelli certificati di inquinanti, con quel po’ di diossina che magari dà quel sapore in più al broccolo, per esempio.

che si traduce in circa 3.500 milligrammi sul secco. Pensate che 1.001 è il limite oltre il quale non si può andare in una discarica ordinaria, ma si deve andare in una discarica per rifiuti speciali pericolosi.

gli interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova; la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti; gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola, Forio, Lacco le misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e 2017. Come già ribadito dal ministro delle infrastrutture Toninelli, con la conversione in legge del decreto ci saranno misure a sostegno delle imprese che hanno avuto difficoltà economiche a causa del crollo, norme che riguardano la zona portuale e retroportuale e aiuti e sostegni anche sul fronte della tassazione ai cittadini che hanno perso la casa a causa del disastro derivante dal crollo del ponte. Vengono disposte risorse per il trasporto locale e per gli autotrasportatori colpiti dalla frattura della viabilità. Non posso quindi negare che sia stato fatto un ottimo lavoro dal nostro Governo e dalla nostra maggioranza, soprattutto alla Camera, dove l’elevata qualità del contributo fornito da ciascuna forza politica ha consentito un lavoro a tratti innegabilmente faticoso, ma estremamente produttivo e di notevole miglioramento del testo. Mi riferisco evidentemente ai significativi interventi per la città di Genova. Non posso, però, non evidenziare la vicenda relativa all’articolo 41, che mi ha visto particolarmente impegnato, anche all’interno del mio Gruppo, a illustrare

Anzitutto, il tema dei fanghi, per la sua complessità e delicatezza, è un po’ estraneo alla questione e mi preme evidenziare una perplessità sull’articolo 41 rispetto alla tutela della salute, che è uno dei nostri princìpi e diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta costituzionale. Mi sono sempre battuto affinché, di fronte alla tutela della salute e dell’ambiente, il profitto potesse fare un passo indietro indietro e ad alcuni di noi sembra che questa norma possa agevolare i profitti di alcune imprese, facendo spandere questi prodotti e queste sostanze sui suoli. Il bene della vita, infatti, merita tutela e l’innalzamento dei limiti di idrocarburi pesanti potrebbe rappresentare un rischio per l’ambiente e per la catena alimentare. È la stessa Unione europea, del resto, che, con le sue direttive, ci invita alla prudenza e a disciplinare l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo. La terra è sacra e non deve diventare una discarica a cielo aperto: dobbiamo preservarla soprattutto per le nostre generazioni future. Sembrerebbe, invece, con il testo pervenuto dalla Camera, di essere di fronte a un aumento dei limiti che, rapportato a quello dei fanghi industriali, è notevolmente superiore. Per queste considerazioni, l’Unione europea ha sempre osservato il principio di precauzione, perché da trent’anni proprio l’Organizzazione mondiale della sanità stabilisce che

Paese. Spero vivamente, quindi, anche alla luce di quanto previsto dal principio di precauzione, che vengano effettuate qui in Assemblea, al Senato, possibili correzioni, al fine di evitare la distribuzione di queste sostanze nei nostri terreni. Chiedo

che ha citato un emendamento del Partito Democratico, riferito al decreto-legge terremoto dello scorso luglio, che tutti insieme abbiamo votato. È stato un riferimento scorretto e per questo intervengo, perché in quest’Assemblea

Altre parti sono state inserite, a nostro avviso malamente; ad esempio, è stata inserita una parte che riguarda anche il Centro Italia. Io sono residente nel cratere di quel terribile terremoto del 2006 bene gli sforzi che abbiamo compiuto; so bene quanti sforzi abbiamo fatto tutti insieme. Ad esempio, colleghi, tutti insieme, a luglio, decidemmo di approvare, in quel provvedimento, che fu l’ultimo atto sulla spinta del Governo Gentiloni Silveri, una sanatoria per le cosiddette piccole difformità. Oggi si fa una cosa molto differente e quando viene citato un nostro emendamento di allora - che tra l’altro non venne votato, perché precluso da quell’accordo che tutti insieme facemmo - viene fatto in maniera

ad esempio il fatto che possano accedere ai contributi solamente i volumi regolarmente accatastati. I limiti sono quelli che stabiliscono che la sanatoria può valere solamente per le piccole difformità e, quindi, relativamente alle percentuali previste dal Piano casa, che nel caso della Regione Marche sono del 20 per cento. Questo limite voi voi di Lega e 5 Stelle lo togliete, permettendo che si vada oltre il 20 per cento e trasformando quella necessità di una sanatoria per piccole difformità in un vero e proprio condono. Voi cancellate il vincolo che noi abbiamo messo e cioè che fossero dei tecnici professionisti ad accertare che non ci fosse un legame tra le volumetrie fatte in maniera abusiva e i danni sismici, perché l’abusivismo causa danni e causa morte, come abbiamo visto nella tragedia che è avvenuta a Palermo.

alle regole (che sono identità) e a un comportamento etico (che è identità) quei vincoli mai li hanno superati. Oggi abbiamo un paesaggio che ci è invidiato in tutta Italia, in Europa e nel mondo. Questi vincoli,

un condono per Ischia che, non a caso, essendo il collegio elettorale del Vice Presidente, è stato chiamato condono Di Maio. Avete inserito delle norme sui fanghi tossici che colpiscono la possibilità di fare agricoltura e la qualità del nostro vivere. Voi ci avvelenate per decreto, Con questo vostro decreto-legge, in cui malamente avete voluto anche inserire queste norme sul Centro Italia, avete cancellato la possibilità

con il crollo del ponte Morandi lo scorso 14 agosto, data di cui oggi ricorrono i tre mesi. Il crollo del ponte Morandi rappresenta il più grave incidente stradale avvenuto nel nostro Paese: grave per il numero di vittime, 43 e che qui voglio ricordare con un sentimento di cordoglio alle famiglie, e per il numero di sfollati, che sono 600, con una sofferenza inflitta a tantissime famiglie. anche per l’importanza della struttura crollata, per l’entità del crollo e per le responsabilità che evidentemente presiedono al disastro, oltre che per l’impatto sociale ed economico sul sistema che ruota attorno alla città di Genova,

Di fronte all’emergenza e alle vittime, le decisioni vengono prese in uno spirito condiviso, perché l’importanza e l’oggettività delle misure da adottare e degli accertamenti da compiere lo consentono e lo pretendono. Noi ci siamo messi, con la nostra parte, a disposizione a tutti i livelli, in più occasioni e a più riprese, ma questo spirito di condivisione, in relazione a questo questo provvedimento e al dibattito che lo ha preceduto, non c’è stato. Non c’è stato per calcolo politico, ma anche per inadeguatezza di questo Governo: un’evidente incapacità ma anche per calcolo politico. Invece di gestire questa crisi con gli strumenti del diritto e della politica a disposizione di chi ha la responsabilità istituzionale, avete scelto una volta di più la via della demagogia, della semplificazione e del pressappochismo, con una serie di annunci vari. Abbiamo avuto un esempio del vostro comportamento nelle settimane e nei mesi successivi annunci di revoca delle concessioni mai attuate, annunci di nazionalizzazioni, nomina di una commissione ispettiva con immediate revoche e dimissioni dei componenti, bozze del decreto-legge senza cifre, dichiarato perfetto in esordio e poi, fortunatamente, in parte modificato. Basti pensare che

Certo, i genovesi si sono rimboccati le maniche, ma da sola Genova non ce la fa. Ed è stato incoraggiante, invece, che la società di civile, le istituzioni, le associazioni anche le forze politiche locali abbiano trovato una capacità di collaborazione e una forza propositiva comune nel chiedere al Parlamento e alla politica la ricostruzione e una risposta a tutte le necessità scaturite dal crollo. Ma, cari colleghi, questo provvedimento è un insieme di soluzioni incomplete, insufficienti e slegate l’una dall’altra. Sono passati tre mesi dal 14 agosto e la città di Genova, considerata anche la la strategicità del Capoluogo ligure dal punto di vista dei transiti commerciali nazionali e internazionali, con questo decreto-legge non ha risposte adeguate. Innanzitutto, non sappiamo chi farà il ponte e quando verrà realizzato. Ci sono annunci vari sui tempi tali da far rabbrividire, per la superficialità con cui viene gestita questa questione, che è dirimente per la sopravvivenza e per il futuro di Genova e della Liguria. L’impalcatura giuridica della ricostruzione è debolissima, come ha detto bene il senatore Margiotta nella sua relazione di minoranza, con un percorso che riteniamo complicatissimo. Non c’è chiarezza sulla ricostruzione, con un’incertezza preoccupante

ma a causa della debolezza giuridica del documento, l’erogazione delle risorse rischia di essere ritardata, se non compromessa, dai ricorsi.

dal punto di vista del sostegno economico e dal punto di vista della progettazione del sistema logistico infrastrutturale: non si parla di Gronda, non si parla di terzo valico e, anche sui risarcimenti alle aziende, il decreto è, ancora una volta, drammaticamente insufficiente. La Camera di Commercio ha stimato un danno per le imprese pari di euro e l’Esecutivo ha stanziato solo delle briciole, perché c’è tutta la parte della zona arancione, dove vi sono aziende e cittadini che stanno soffrendo in via indiretta. E sono briciole anche quelle messe per il porto di Genova. Noi abbiamo proposto la Zona economica speciale, che è anche una misura di sviluppo, ma non è stata presa in considerazione. Il decretolegge non contiene inoltre alcuna misura soddisfacente per la zona franca, per la cassa in deroga. Vorrei spendere qualche parola sulle grandi opere, perché l’isolamento che Genova sta vivendo, e rischia di vivere ancora a lungo, dovrebbe far comprendere a tutti l’importanza strategica della Gronda e del Terzo valico. E invece, proprio nella discussione di questo provvedimento, abbiamo dovuto sopportare i soliti preconcetti ancorati all’idea della decrescita felice.

la nostra amata Genova ha subìto uno dei fatti più tragici della recente storia repubblicana, una sciagura che ha cause lontane perché da anni, appunto, il Paese risente di un’incuranza, di una cattiva gestione della cosa pubblica, dell’illegalità diffusa, connivenza tra parte peggiore dell’imprenditoria e apparati pubblici che non svolgono la funzione e i compiti per i quali sono preposti. Al di là delle responsabilità civili e penali che verranno accertate, non possiamo esimerci dall’affermare che quello che è accaduto sia lo specchio del malsistema che ha caratterizzato l’Italia negli ultimi decenni, quello che stiamo combattendo

nostro esame non si limita, però, ad affrontare solo la grave situazione del crollo del ponte di Genova, quindi quella emergenza. In qualità di componente della Commissione lavoro, e insieme ai miei colleghi della Commissione, vogliamo esprimere in questa Aula la nostra massima soddisfazione per come il provvedimento interviene proprio in materia di lavoro. Tra le misure più importanti, infatti, c’è anche la reintroduzione della cassa integrazione per cessazione.

si sono trovati a rischio licenziamento a causa della scadenza della cassa integrazione per cessazione, non più rinnovabile proprio per le limitazioni imposte dalla riforma del lavoro del Governo Renzi. Con gli effetti del decreto, i lavoratori potranno ritornare ad usufruire della cassa integrazione per un massimo di dodici mesi per gli anni 20192020, riuscendo così a riordinare la propria vita e ad adoperarsi con maggiore tranquillità per trovare un nuovo lavoro. Siamo in un momento particolarmente difficile per il mondo del lavoro: la crisi economica si somma alle problematiche relative alla delocalizzazione aziendale, a causa delle aziende che trasferiscono le loro produzioni all’estero, chiudendo stabilimenti storici. gli ammortizzatori sociali proprio in questo momento, da parte del precedente Governo, è stato veramente un atto allucinante e improponibile. Come maggioranza, in questi primi mesi di legislatura, insieme al ministro Di Maio, siamo impegnati in numerosi tavoli di crisi, uniti nell’intento di difendere i diritti dei lavoratori per migliaia di nostri concittadini. Personalmente, sono stato orgoglioso di partecipare al tavolo che

riforma sulla cassa integrazione per cessazione, non perderanno il proprio lavoro e potranno rientrare nel tessuto produttivo. Con orgoglio, quindi, e ad alta voce, possiamo confermare, come ha sostenuto il nostro ministro Di Maio, che questo è un Governo che non abbandona le persone. Ecco cosa spinge la nostra azione all’interno delle istituzioni, questo è il vero cambiamento: dopo anni di totale disinteresse, lo Stato torna finalmente a fare lo Stato. (Applausi dal

Signor Presidente, colleghi, rappresen- tanti del Governo, ai colleghi del Partito Democratico, che accusano questa maggioranza di aver fatto poco per Genova e una schifezza per Ischia, dico che sono ipocriti e in malafede. Nel decreto-legge a Ischia sono dedicati 20 articoli, con misure strutturali per affrontare seriamente il post-emergenza e la ricostruzione. Mi rivolgo alla collega Valente - che non vedo della conversione del decreto-legge n. 55 si era scagliata contro la nuova maggioranza, perché non aveva previsto misure per le comunità ischitane: queste misure sono le risposte al nulla del Governo Gentiloni Quello che c’è nell’articolo 25 non è un nuovo condono né un condono tombale. L’articolo 25, che avete preso di mira, ambisce solo a chiudere domande ancora aperte relative a condoni precedenti. Dite che ne beneficeranno tutti i 28.000 edifici abusivi dell’isola di Ischia: è un falso. Si affronteranno solo domande relative a edifici distrutti o danneggiati dal dal terremoto del 21 agosto 2017 e di soli tre Comuni dell’isola (Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno). Stiamo parlando dunque di meno di un migliaio di edifici e preciso che nessun condono ci sarà per chi è stato condannato per criminalità organizzata o riciclaggio e sarà necessaria l’autorizzazione paesaggistica. dunque, dove ci sono vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici e archeologici. Non ci saranno dunque condoni per edifici costruiti in alvei o nei pressi di torrenti o fiumi. Non ci saranno dunque condoni per case costruite su versanti franosi o dove ci sono vincoli di inedificabilità assoluta. Nessun contributo per volumi oggetto di condono. Certo, l’articolo 25, com’è stato emanato dal Governo, presentava qualche criticità, ma noi della Lega - e lo rivendichiamo - lo abbiamo migliorato. Voi delle opposizioni siete così poveri di argomenti che tentate di gettare fango ovunque (a proposito di fanghi da depurazione). Ci accusate anche di aver introdotto una sanatoria grave

per sbloccare e accelerare la ricostruzione ancora ferma al palo per vostra incapacità e responsabilità. (Applausi dai Gruppi L- SP-PSd’Az e M5S). Cosa abbiamo fatto di tanto grave? Semplice, abbiamo uniformato in tutti i territori del cratere le procedure già previste in due Regioni.

dove, con legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, avete previsto le sanatorie di non conformità. Dunque, voi del Partito Democratico, con leggi regionali, avete già previsto di sanare in non conformità.

Abbiamo riconosciuto il ruolo fondamentale dei Comuni nella cabina di regia del commissario; le università diventano soggetti attuatori sui propri immobili danneggiati; vengono ampliate le misure per intervenire sulle 3.000 chiese distrutte o danneggiate. Per noi la fruibilità di questi luoghi di culto è fondamentale per le comunità colpite. inoltre prevista la definitiva delocalizzazione delle stalle collocate in strutture temporanee, fondamentale per le imprese agricole. Viene anche prevista l’anticipazione dei compensi

questi poteri fondamentali per accelerare i lavori e l’ottenimento delle autorizzazioni, ma non dimentichiamo i problemi che stanno gravando sui

lasciando agli altri amici del Gruppo la trattazione di temi di contenuto diverso all’interno del decreto-legge.

presidente, onorevole Bernini, abbiamo più volte chiesto al Governo un provvedimento specifico per il terremoto di Ischia, che per noi rappresenta una vera e propria emergenza alla quale bisogna dare risposte. Il Gruppo Forza Italia è stato chiaro sul punto fin dall’inizio; lo abbiamo sempre sostenuto e prendiamo atto che all’interno del decreto-legge il Governo ha dedicato uno spazio importante alla trattazione dei problemi che riguardano l’isola di Ischia.

chi dovrebbe vergognarsi sono gli esponenti del Partito Democratico ai massimi livelli, fino ai rappresentanti locali, che non hanno avvertito un senso di dignità messi in una posizione diversa rispetto ai loro vertici nazionali, lasciando che sul territorio si dicesse una cosa e ai vertici nazionali un’altra.

dalla Sicilia alle Alpi: vive forse qualche problema di natura diversa ma non si differenzia dalle altre. Ci sono sull’isola d’Ischia, come in molti territori della Regione Campania, cittadini che, non per colpa loro ma per colpa della mancanza di risposte della politica negli ultimi trent’anni, vivono un momento di grossa difficoltà.

nel suo contenuto? Si «definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017». Questo è il testo originale dell’articolo 25. I Comuni danneggiati dell’isola d’Ischia sono il Comune di Casamicciola Terme, il Comune di Lacco Ameno e il Comune di Forio. Questi tre Comuni,

nostro esame presenta certamente delle risposte importanti e ha dei contenuti positivi. Si dà la possibilità di accelerare l’esame delle pratiche di condono

i vincoli assolutamente inderogabili. Non si può costruire sul ciglio della strada e, quindi, non si può rilasciare concessione in sanatoria: se c’è una costruzione abusiva sul ciglio della strada, va abbattuta. Non si può costruire e sanare vicino a un bene di pregio dal punto di vista archeologico: non è possibile; lo stabilisce la norma.

hanno necessità di alcune risposte. Prendiamo atto con soddisfazione che in questo Parlamento si inizia a parlare finalmente, in maniera costruttiva, di un tema che coinvolge tante comunità

Trovo anche doveroso iniziare questo mio intervento con un ricordo delle 43 vittime che hanno perso la vita il 14 agosto. non siano in questo momento presenti in Aula e, appunto, mi rammarico del fatto che, come avvenuto in Commissione, appena finiti i loro interventi abbiano lasciato le loro posizioni. Ma comunque andrò avanti. Il crollo del Morandi, con i suoi 43 morti, i feriti, gli sfollati, gli immani danni e disagi che quotidianamente stiamo subendo noi genovesi,

Il crollo del Morandi, con i suoi 43 morti, i feriti, gli sfollati, gli immani danni e disagi che quotidianamente stiamo subendo noi genovesi, non è un caso isolato: è solo l’ultimo ed il più grave episodio di una serie impressionante di cedimenti delle nostre infrastrutture. Si può dire che non vi sia stato uno solo degli ultimi cinque anni in cui almeno un ponte, un cavalcavia non sia crollato da qualche parte della nostra Penisola. Nel 2013 a Carasco, sempre vicino a Genova, vi fu il crollo di un ponte che uccise due persone. Nello stesso anno crollarono anche un ponte in Sardegna e un viadotto in Sicilia.

Ad ogni crollo, morti, feriti e ingenti danni. La precaria situazione delle nostre infrastrutture deve inoltre fare i conti con la fragilità del nostro territorio, che ogni anno frana o si allaga sotto i colpi di eventi atmosferici estremi che si ripetono con sempre maggiore frequenza. Ne è un triste esempio l’ondata di maltempo che si è susseguita dall’inizio di ottobre provocando ancora crolli, ancora disastri, ancora esondazioni da Nord a Sud. al cospetto di tali macerie, quali ulteriori prove ci occorrono per comprendere che, se non interveniamo immediatamente, le nostre infrastrutture collasseranno con ancora maggiore frequenza, le nostre strade franeranno e i nostri quartieri continueranno ad allagarsi? Quali altri segnali dobbiamo attendere per comprendere che l’urgenza non sono le nuove grandi opere, ma la manutenzione e la messa in sicurezza delle opere che già abbiamo? Ogni centesimo che noi sottrarremo alla prevenzione e alla messa in sicurezza delle nostre infrastrutture e del nostro territorio ci costringerà a piangere ancora morti e a contare ancora danni. Il decreto-legge che oggi siamo chiamati a convertire ci dimostra due cose. La prima è che porre rimedio ai danni provocati dall’incuria su opere e territorio è assai più costoso che prevenire tali danni. La seconda è che il Governo e questa maggioranza hanno ben chiaro che la prevenzione è l’investimento migliore e più remunerativo che possiamo mettere in atto. Sotto il primo profilo, cioè per l’emergenza Genova, mi limiterò a descrivere per sommi capi lo sforzo immane di energie e risorse che questo Governo, a partire dal 14 agosto, ha dovuto compiere. Il 15 agosto il Presidente del Consiglio, recatosi immediatamente a Genova insieme al vice premier Di Maio e al ministro Toninelli (io ero presente) ha annunciato il primo stanziamento di cinque milioni di euro per far fronte alle necessità più urgenti, divenuti oltre 33 con il Consiglio dei Ministri del 18 agosto ed aumentati dal decreto che ci accingiamo a convertire di ulteriori nove milioni per il 2018 e 11 milioni per il 2019. Il 20 agosto Genova già poteva contare, oltre che sui primi stanziamenti economici, anche sullo strumento giuridico con cui il commissario delegato all’emergenza ha potuto operare per tentare di garantire la ripresa delle normali condizioni di vita dei genovesi. Il 28 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di cui discutiamo oggi, che ha previsto la nomina del commissario straordinario per la ricostruzione. Nell’ultimo mese in Parlamento, insieme ai miei colleghi, abbiamo lavorato incessantemente, senza conferenze stampa o proclami, ma in silenzio e a testa bassa - come piace a noi genovesi - ascoltando minuziosamente tutti i soggetti coinvolti, che hanno dato consigli e anche fatto critiche utili a migliorare questo decreto. Grazie a questi sforzi, il commissario per la ricostruzione potrà operare velocemente in deroga ad ogni disposizione di legge (salvo quella penale e al codice antimafia), coadiuvato da una struttura per la quale è stata autorizzata la spesa di 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

pur dovendo far fronte alle spese di ricostruzione. In caso di mancato o ritardato pagamento, il commissario individuerà un soggetto che anticiperà le somme a fronte della cessione del credito, garantita con uno stanziamento di 30 milioni annui dall’anno 2018 all’anno 2029. Più di 72 milioni di euro verranno assegnati alle famiglie degli sfollati; più di 15 milioni di euro sono stanziati per assumere personale a supporto dell’emergenza negli enti locali, nell’Autorità di sistema portuale, negli uffici giudiziari, nell’Agenzia delle dogane e nella Direzione marittima; 55 milioni verranno impiegati a supporto delle imprese, le quali potranno beneficiare della semplificazione amministrativa prevista dalla zona logistica semplificata, nonché degli sgravi introdotti dall’istituzione della zona franca urbana. Sono inoltre previsti 30 milioni per sostenere i lavoratori dipendenti e autonomi; a sostegno del trasporto pubblico locale sono stanziati più di 43 milioni, oltre a 20 milioni per il rinnovo del parco mezzi, con priorità per quelli a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno; 20 milioni sono stanziati per gli indennizzi agli autotrasportatori. Si prevede inoltre la progettazione e la realizzazione di infrastrutture di alta automazione per garantire l’ottimizzazione dei flussi veicolari in ingresso e in uscita dal porto, con autorizzazione alla spesa di 30 milioni; 45 milioni vengono stanziati affinché il porto di Genova non perda i suoi traffici e per incentivare il trasporto delle merci su rotaia (il cosiddetto ferrobonus). Ma lo vedete quante energie e quante risorse il Governo e questa maggioranza hanno profuso? In tutto nei prossimi tre anni Genova potrà contare su più di 700 milioni per tentare di non scivolare nel declino che il crollo del Morandi potrebbe provocare. Il decreto-legge in questione, tuttavia, non si limita a fare tutto quanto è possibile per Genova, ma dimostra che questo Governo intende invertire la tendenza in fatto di prevenzione e sicurezza. Il decreto-legge infatti sancisce finalmente che, entro dodici mesi, tutte le concessionarie autostradali debbano verificare e mettere in sicurezza le infrastrutture viarie loro affidate, senza poter aumentare le tariffe. Di straordinaria importanza è poi l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, che avrà il compito di controllare e verificare quello che i concessionari faranno, garantendo così la sicurezza delle nostre infrastrutture; per fare ciò, potrà assumere più di 209 dipendenti, Con il decreto-legge in conversione, inoltre, viene istituito l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche in cui confluiranno tutti i dati tecnici, amministrativi, di gestione e di efficienza di ponti, viadotti, cavalcavia (sia stradali che ferroviari), porti, aeroporti, dighe, gallerie, infrastrutture ed edifici pubblici. Sempre nell’ottica della prevenzione, viene poi progettata la realizzazione di un sistema di monitoraggio dinamico, con uno stanziamento di 15 milioni. Si prevede infine un piano di monitoraggio e conservazione dei beni culturali, con stanziamento di altri 20 milioni. Per realizzare tali obiettivi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nel 2019, 200 unità di personale, prevalen di più 7 milioni annui a decorrere dal 2019. Lo sforzo economico messo in campo è enorme e il cambio di passo è evidente: da una cultura dell’emergenza finalmente si tenta di passare a una cultura della prevenzione. Per tutti questi motivi il mio giudizio non può che essere positivo. Per questi motivi voterò a favore della conversione del decreto-legge, con la convinzione di contribuire, oltre che a porre rimedio ai danni provocati alla mia città, anche allo sforzo di riedificare uno Stato dalle rovine materiali e morali che ci avete lasciato.

una viabilità sotto il viadotto, è stata aperta ex novo una viabilità portuale, è stato anticipato un cantiere di collegamento tra autostradale di Genova Aeroporto e Genova Ovest, che doveva terminare a giugno o luglio del prossimo anno e invece verrà terminato a novembre di quest’anno per le prime due corsie e il resto verrà realizzato entro febbraio del 2019. Questo per dire che in realtà, oltre ad aver dato la possibilità agli sfollati di poter tornare, in sicurezza, a prendere i propri beni all’interno delle case, anche per questa operazione, non solo tecnicamente difficile ma anche chiaramente onerosa, il Governo ha proceduto a coprire integralmente i costi. Lo dico perché ad onor del vero vi è stata grande collaborazione con le amministrazioni locali, con il commissario delegato per l’emergenza - il presidente Toti - e con

14 Novembre 2018 quanto stabilito nella manovra che prevede ulteriori risorse stanziate per l’evento e che porterà ad un ammontare complessivo di oltre un miliardo di euro per l’area genovese e ligure e soprattutto per la capacità logistica del primo scalo italiano. Quindi non si tratta di un decreto che non stabilisce delle misure: è un decreto che, per chi come me è di quel territorio e ne conosce

Detto questo, si poteva far meglio? Sì, si può sempre far meglio e si può sempre migliorare. Credo però che il benaltrismo non aiuti a risollevare la situazione di una città che ancora vive il disagio profondo di essere tagliata in due e di una catena logistica e industriale italiana del Nord-Ovest che ha grandissime problematiche quando il primo scalo del Paese va in forte sofferenza. Quindi credo che se nella giornata di oggi - o domani mattina - il Senato della Repubblica contribuirà con la sua azione a convertire in legge questo decreto darà darà un aiuto concreto alla città, alle aziende, ai lavoratori che aspettano delle risposte con la cassa integrazione in deroga e a tutte quelle realtà che in questi mesi, seppure con sofferenza, non si sono fermate e hanno continuato a operare a Genova portando avanti importanti pezzi della ricostruzione, che non inizierà domani perché è iniziata ieri. Domani noi contribuiremo, se convertiremo in legge questo decreto, a dare gli strumenti al commissario straordinario per poter immediatamente procedere all’assegnazione dei progetti e all’assegnazione del cantiere. Questo è lo scopo del decreto che non è l’unica soluzione di fronte a un problema che ha sconvolto il sistema logistico italiano ma è uno degli strumenti che noi mettiamo a disposizione per riuscire a risollevare rapidamente l’economia di una parte importante di questo Paese. Questi sono dunque

che non sono incerti, come dice qualcuno, ma attendono una risposta da questa Camera, affinché si possano avere gli strumenti necessari a far partire finalmente i lavori di demolizione e di costruzione del viadotto. Senza questo via libera,

nello svolgere un ruolo che in questo momento è fondamentale per rilasciare un territorio come quello di Genova, della Liguria e dell’intero Nord-Ovest del Paese.

Oltre a tutte le misure a sostegno di Genova elencate adesso dal collega Rixi, è prevista sempre su Genova - ma non solo per Genova - l’assunzione straordinaria di 50 unità al Ministero della giustizia:

la nomina di un Commissario straordinario per il terremoto di Ischia, che potrà vigilare e coordinare le operazioni di ricostruzione al fine di ridurre i rischi sismici, idrogeologici e occuparsi della tutela paesaggistica. Dopo questi interventi 1.000 edifici saranno più sicuri: questo è il dato di fatto. poi l’accertamento e il recupero delle risorse per il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici per rimodulare la destinazione delle scuole entro il 2018, quindi la messa in sicurezza delle scuole. semplificazione delle procedure per il sisma del Centro Italia. Parliamoci chiaro: oggi ci sono alcune Regioni del Centro Italia nelle quali è consentito, dalle relative leggi, di poter richiedere un ampliamento della volumetria; è consentito dalle leggi regionali.

ciò che è consentito dalla legge regionale si fa contestualmente alla domanda del contributo per la ricostruzione. contributo di 2 milioni di euro per la riapertura del viadotto Sente, altra struttura bloccata. Vi è lo sblocco delle risorse per gli interventi di messa in sicurezza dell’autostrada dei parchi A24-A25, anticipando subito 250 milioni di euro. Si stanziano 9 milioni di euro per ciascuno dei tre anni successivi per la progettazione delle scuole innovative e dei poli dell’infanzia. È stato introdotto, con l’articolo 44, il trattamento di integrazione salariale per le imprese in crisi, che ha reso possibile salvaguardare il reddito dei lavoratori delle imprese che sono in crisi, che stanno cessando l’attività o che hanno concrete prospettive di cederla

trent’anni perché un Governo finalmente (evidenzio questa parola: finalmente), sebbene per una fase transitoria, mettesse un limite allo spandimento dei fanghi.

alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Su questo c’è l’impegno del Governo a rivedere in maniera organica tutta la normativa, non solo sui fanghi, ma anche sui gessi di defecazione, che sono un derivato dei fanghi.

ma oggi credo che tutti abbiamo preso coscienza del perché questo è il Governo del cambiamento. C’è proprio la rappresentazione fisica del Governo del cambiamento, perché ci eravamo abituati in Aula, sia alla Camera che al Senato, al fatto che dopo la discussione replicassero un esponente della maggioranza e uno del Governo. Invece, con il Governo del cambiamento, abbiamo due esponenti che intervengono come Governo. Grazie per questa illuminazione che da oggi ho compreso.

Benissimo,

Signor Presidente, intervengo perché in queste set- timane, soprattutto in Commissione, chi ha partecipato ai lavori si è impratichito su delle zone: si parla della zona rossa e si è parlato della zona arancione. La zona rossa è quella immediatamente colpita dal fenomeno, ma chiunque abbia un’idea di Genova sa che quel crollo è stata una ferita che ha riguardato tutta la città. Divide sulla traiettoria Ovest-Est ma anche NordSud e via Walter Fillak, che è quella via che unisce Sampierdarena e Certosa, è di fatto bloccata e quello che era un percorso normale, cioè poter attraversare una via per arrivare da un quartiere

come è stato giusto fare, agli sfollati della zona rossa, ma anche alla zona arancione. È assolutamente essenziale. Pensate che abbiamo tenuto un’assemblea in Valpolcevera per sentire le varie esigenze e un lavoratore ci ha raccontato come

che hanno partecipato a questa assemblea, hanno detto che nel decreto hanno trovato rispondenza su molte cose ma che si preoccupano perché sta morendo tutto il tessuto dentro il quale sono vissuti. Vi chiedo quindi veramente di cercare di votare a favore di questo emendamento, perché non è una richiesta solo del PD, ma di tutta la comunità genovese.

Guardo lui e guardo il ministro Toninelli; esprimo tutta la mia solidarietà al vice ministro Rixi, perché so che su questo ordine del giorno la pensa come noi: lo ha detto più volte, anche in interviste.

porta a una decisione totalmente politica. Il costo iniziale, ma soprattutto quello finale, è un numero. Il beneficio invece non è un numero, il beneficio non è solo economicista, ma viene valutato sulla base della propria sensibilità culturale. Ad esempio, per un Governo fare un campetto di calcio in un piccolissimo paese è uno spreco, mentre per un altro spendere soldi per l’integrazione degli immigrati è invece una cosa vantaggiosa. Ho fatto questi esempi solo per dire che ha ragione l’esperto che avete nominato, che dice che essi faranno le loro valutazioni, ma che alla fine deciderà la politica. Allora, la politica, che è qui nelle sue massime espressioni con il Ministro dei trasporti, ci può dire se il terzo valico lo volete fare oppure no? Ne prenderemo atto. Ci vuole un po’ di serietà e di assunzione di responsabilità. L’ordine del giorno dice solo: lo vogliamo fare?

Signor Presidente, mi stupisco molto di questo parere contrario senza neanche un tentativo di modifica dell’ordine del giorno, perché forse il Governo poteva - per esempio - accettare almeno il primo impegno: «considerata la straordinarietà della situazione (…) sbloccare le risorse relative al V Lotto». Dico questo perché nelle dichiarazioni del Governo è stato detto che le risorse approvate dal CIPE a luglio ci sono

un tale imbarazzo nel Governo che, quando si parla di Terzo valico, non si accoglie neppure quella parte che si è detto già esserci? È grave. grave, e qui mi ricollego alla città, perché chiunque conosca la città di Genova sa che il problema della circolazione non è soltanto conseguente al crollo del ponte Morandi. Chi percorreva quel ponte faceva spesso ore di coda per arrivare da ponente al porto, perché su quel ponte passavano i TIR; su quel ponte passava il traffico cittadino; su quel ponte passavano coloro che dovevano transitare da Genova e a Genova non si dovevano fermare. Allora, per una grande città come Genova, per il più grande porto del Mediterraneo la cui vocazione è permettere di entrare e uscire, il futuro e lo sviluppo sono connessi a questo: non si può fare a meno di quest’opera. Davvero mi colpisce che sia stato dato parere contrario senza neppure

approva. (v. Allegato B). Onorevoli colleghi, in conformità a quanto già stabilito durante l’esame in sede referente, la Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 4.11

Dichiara altresì inammissibili gli emendamenti 3.12 e 5.14, in quanto privi di portata modificativa, nonché la proposta 41.18, che reca una delega senza l’indicazione di principi e criteri direttivi.

PRESIDENTE. Siamo lieti di salutare gli studenti dell’Istituto di istruzione superiore «Alfredo Panzini» di Senigallia, che assistono ai nostri lavori.

stiamo votando una serie di e- mendamenti presentati dal Partito Democratico che riguardano il sostegno ai lavoratori che, a seguito del crollo del ponte Morandi, stanno vivendo una situazione di estrema difficoltà. Mi riferisco sia ai lavoratori che hanno dirit in deroga, sia a quelli per cui sono necessari altri tipi di supporti perché non sono coperti da questo ammortizzatore sociale. L’intervento che è stato proposto dal Governo in tal senso

che le lentezze sono dovute all’opposizione che fa ostruzionismo. Qui nessuno ha fatto ostruzionismo, ma - anzi - abbiamo cercato di migliorare il testo. I tempi lunghi sono tutta responsabilità del Governo. Per i lavoratori che soffri-_ ranno anche di questi tempi lunghi, che sono vostra responsabilità, noi chiediamo che ci siano più risorse e più tempo per reperirle.

circa due mesi fa, subito dopo i tragici eventi del ponte Morandi, in quanto tutta la rete stradale della provincia di Alessandria è sottoposta

l’emendamento in questione si riferisce a una parte delle grandi infrastrutture che interessano la realtà genovese, in particolare il Terzo Valico dei Giovi. Noi poniamo l’attenzione su questa infrastruttura, perché non condividiamo nella maniera più assoluta

quella portuale, quella aeroportuale, quella del futuro della città, che potrebbe incidere molto negativamente sullo sviluppo e sulla crescita. Quindi noi poniamo all’attenzione dell’Assemblea la necessità che si prosegua nella progettazione e nella parte esecutiva del Terzo Valico, perché lo riteniamo parte fondamentale per la crescita della Liguria e di Genova in particolare.

conforme al relatore.

Signor Presidente, l’articolo 7 istituisce la Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto di Genova, fino ad includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzo e Melzo e Vado Ligure. Essere inclusi nella zona semplificata consente alle imprese del settore, operanti su questi siti, il beneficio di godere di procedure semplificate e, conseguentemente, minor costi, maggiore competitività, possibilità di beneficiare di contributi pubblici. Restano esclusi l’interporto di Torino Orbassano, Mondovì e Novara, quest’ultima collocata proprio sulla direttrice GenovaMilano.

alle città che rimarranno escluse dalla zona logistica. Allora mi chiedo perché non farlo nella sede opportuna, qui in Parlamento?

avendo la facoltà fino all’ultimo momento di concedere l’opzione dell’integrazione in questo elenco. Se le intenzioni sono davvero quelle di ampliare la zona logistica semplificata, perché non approvare il nostro emendamento, che integra e amplia la lista dei retroporti di Genova, includendo appunto le città importanti di Torino, Orbassano, Mondovì e Novara.

abbiamo chiesto di attivare un tavolo istituzionale anche per la zona logistica di La Spezia e per il retroporto di Santo Stefano Magra. Su un analogo ordine del giorno alla Camera dei deputati c’è stata una sorta di condivisione

l’attuazione delle norme previste da questo decreto-legge, per verificare l’opportunità di estendere i periodi, in quanto l’indicazione specifica di un’estensione del periodo di calcolo del fatturato che ha subito un decremento potrebbe anche avere degli effetti negativi nei confronti delle imprese che possono accedere a questo contributo.

conforme al relatore.

Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché, come ricordavo prima, questo decreto-legge ha avuto una serie di versioni. Una prima versione, prima che passasse in Consiglio dei Ministri, aveva significative significative risorse per il porto di Genova. Vedete, il porto di Genova è, di fatto, il più grande datore di lavoro del Nord-Ovest (si parla di 176.000 addetti, fra diretti e indiretti), quindi non è importante solo per Genova, ma per l’Italia intera. Chi lavora in porto sta verificando che, già adesso, c’è un 20 per cento di entrate in meno di tasse portuali rispetto a quello che succedeva prima del crollo del ponte Morandi. Per non parlare poi dei disagi che hanno gli autotrasportatori: pensate di quanto hanno dovuto allungare il tragitto e quanto costa di più per loro dover portare le merci, non solo in termini di tempo, ma di benzina e di ore lavorate. Soltanto per gli autotrasportatori si è calcolato un danno economico di 6,5-6,6 milioni di euro. Voi capite allora che le risorse che sono state stanziate per il porto sono pochissime rispetto ai danni che sta subendo. Chi lavora in porto dice: dateci almeno la certezza di chi ricostruirà il ponte e in quanto tempo, altrimenti chi si deve organizzare si riorganizza e i traffici, invece che continuare ad arrivare a Genova, vanno da altre parti e neppure d’Italia, ma a Rotterdam o ad Anversa.

Allora, dato che stiamo ragionando contestualmente di manovra di bilancio e di questo decreto-legge, perché non inserire qui un emendamento che dice: diamo le risorse al ponte e poi si troverà nella legge di bilancio la copertura? Se questo non si fa, mi dispiace: allora le promesse, date date a mezzo stampa, di trovare più risorse per il porto di Genova sono promesse vacue. Se le promesse invece vogliono avere qualcosa di scritto e di reale, bisogna votare questo emendamento.

una modifica semantica lessicale: il condono edilizio si può anche chiamare intervento chirurgico, ma sempre condono edilizio è. Si può cambiare il significante, ma il significato rimane sempre lo stesso. Il senatore Castaldi questa mattina ha detto che stanno cercando di fare ciò che non abbiamo fatto noi. Ha capito esattamente lo spirito. Noi non abbiamo mai fatto alcun condono, mentre, come abbiamo già ripetuto e dimostrato questa mattina nella relazione di minoranza, questo è il quarto condono. Il Movimento 5 Stelle lo fa dopo cinque mesi di Governo, la Lega lo fa per la terza volta al terzo Governo a cui partecipa. una nota collegata all’emendamento; nella seduta di Commissione di ieri, Presidente, nessuno del Partito Democratico è uscito. Siamo stati fino alla fine a votare. Ci risulta invece che sia stato cacciato dal Movimento 5 Stelle chi difende la legalità, ma su questo farete voi i conti.

alla Camera, c’è stata una battaglia sul famoso disegno di legge Falanga, che aveva ad oggetto proprio la questione degli abusi e dei condoni in Campania e, in particolare, ad Ischia. Voglio illustrare rapidamente l’emendamento soppressivo per rispondere anche a una serie di questioni e di obiezioni poste

arriverà un condono. Questo è quanto state facendo alla faccia della legalità e dell’onestà.

tende a ripristinare la differenza di regime tra le leggi sul condono edilizio, cioè tra la legge n. 47 del 1985, il condono del 1994 e il condono del 2003. Anche se è condivisibile sul piano teorico dall’esigenza di condurre a una coerenza il sistema normativo, non viene considerata però la specificità dell’ambito in cui la norma emendata è destinata a produrre i propri affetti e ciò non solo e non tanto per la natura emergenziale della previsione dell’articolo 25 del decreto-legge in esame, che nasce con lo scopo di favorire la ricostruzione nei Comuni danneggiati dal terremoto nell’isola d’Ischia, quanto piuttosto per consentire l’effettivo smaltimento delle giacenze delle domande di condono esaminabili solo mediante l’impiego, sia pure in via sussidiaria, dei criteri di valutazione stabilite dalla legge n. Infatti, solo in questo modo potranno essere esaminate le domande relative al condono del 1994 e a quello del 2003, altrimenti non esaminabili, in quanto ancora manca il livello di pianificazione paesaggistica di competenza dell’amministrazione dei beni ambientali. Voglio ricordare a me stesso e a questo Parlamento che la Regione Campania è ancora l’unica Regione in Italia sprovvista di un piano paesaggistico, cioè di una legge che regoli, attraverso le proprie norme, lo sviluppo del territorio e la tutela del paesaggio. Questo non è ancora consentito a noi cittadini campani e di questo dobbiamo ringraziare i governi regionali della sinistra degli ultimi vent’anni.

Infatti, l’articolo 33 della legge n. 47 del 1985 indica in maniera chiara i casi di incondonabilità assoluta e l’articolo 32 quello di condonabilità relativa, nel senso che la pratica è ammessa a sanatoria solo dopo il parere favorevole della soprintendenza. Occorre dunque ripristinare la formulazione originale del primo comma dell’articolo 25 del decreto-legge, che l’emendamento votato ieri in Commissione ha modificato modificandolo produrrebbe, se questa Assemblea conferma il voto di ieri in Commissione, la possibilità che la ricostruzione nei Comuni colpiti dal terremoto dell’isola d’Ischia non avvenga. Per questo chiedo, innanzitutto al mio Gruppo

e anche nel corso della campagna elettorale, non possiamo che votare contro l’articolo 25 e quindi a favore degli emendamenti soppressivi dei singoli commi e dell’articolo. perseguire l’onestà anche nelle parole e nei concetti: tutto quello che aiuta a realizzare o a perfezionare un condono è esso stesso un condono. Questo dobbiamo dircelo chiaramente; non possiamo girare intorno alla realtà. intorno alla realtà. Noi conosciamo la realtà di Ischia, come la conoscete voi, ma la conoscevamo prima, come la conoscevano i colleghi ora al Governo, quando predicavano cose molto diverse,

perlomeno meno impattanti rispetto a quelle scritte in questa norma. Riteniamo che un condono vada perlomeno pagato:

ai cit- tadini di sanare abitazioni, edifici, alberghi, seconde case e Dio solo sa che cosa, senza pagare un solo euro all’amministrazione del Comune o dello Stato, salvo poi finanziare queste stesse persone con i soldi dei cittadini. Avete realizzato un vero capolavoro del rinnovamento della politica: complimenti. Il nostro voto sarà coerentemente contrario a questo provvedimento. (Ap- plausi dal

Questi emendamenti nascono proprio dall’esigenza di chiarire a tutti che il MoVimento 5 Stelle non ha mai inteso e non intende dare vita a un nuovo condono. Siccome nel decreto-legge Siccome nel decreto-legge si dà un termine di sei mesi a tutte quelle domande che sono ad oggi ancora sospese, con questi

perché non estendere a tutti i Comuni d’Italia il termine di sei mesi? Così tra sei mesi avremo la mappa di tutte le case che sono da abbattere e potremo dare vita a questo piano fantastico di demolizione di tutte le case abusive,

vorrei fare un attimo di chiarezza in merito all’articolo 25, approfittando di questa seconda lettura in Senato per chiarire alcune cose. Non c’è nessun potenziamento di condoni. (Commenti dal valutazione preferenziale in termini di tem- pistica, con attività veloci, esclusivamente - ci tengo a precisarlo - per gli edifici danneggiati dal sisma. Ho qui alcuni dati che vorrei leggervi perché è bene che tutti sappiano di che numeri e di che cosa stiamo parlando, prima di parlare di condoni e di condoni tombali.

quelle del 2003, cioè quelle che secondo chi obietta rispetto al contenuto di questa legge avrebbero una corsia preferenziale con una deroga, sono 368: Gruppo PD). Vi chiedo di ascoltarmi fino in fondo, se avete questa correttezza. Io vi ho ascoltato in silenzio come tutti gli altri. per cento del totale. Quanti sono gli immobili danneggiati dal sisma nel Comune di Lacco Ameno?

se la matematica non è un’opinione (e anche la statistica), se il 20 per cento delle domande sono del 2003, posso immaginare che le domande di condono di edifici danneggiati dal sisma

Per poter definire le procedure di contributi per la ricostruzione, ove spettanti, tengo a precisarlo, è necessario

rispetto alle tante falsità che sono state dette in questi giorni. L’articolo 33 della legge n. 47 del 1985 - non 2003 - dice che non potranno essere sanati in alcun modo immobili ubicati in aree sottoposte a vincoli di inedificabilità assoluta e questo già vi da un’ulteriore garanzia. Aggiungo un altro elemento: prima di procedere alla ricostruzione, come sapete, è stato nominato un commissario straordinario che non è un’autorità politica, quindi possono essere mosse critiche alle istituzioni che hanno ritardato trentatré anni per definire le domande di condono presentate a suo tempo, ma il commissario straordinario, d’intesa con la Protezione civile, ha già avviato l’attività di valutazione per la microzonazione sismica e quindi sarà effettuato un piano di delocalizzazione perché le eventuali ricostruzioni, ove spettanti, ove aventi diritto alla ricostruzione e alla contribuzione, avvengano comunque in sicurezza.

mille abitazioni saranno antisismiche, saranno tolte da situazioni di rischio idrogeologico e saranno delocalizzate ai fini della tutela paesaggistica. Questa è ministri. Questo è ciò che accadrà, e il Governo, al termine dei sei mesi, ri- ferirà al Parlamento sullo stato dell’arte.

Presidente, intervengo sulla soppres- sione dell’articolo. Vorrei ricordare al Sottosegretario, che certamente ne è consapevole, che il titolo dell’articolo 25 è: «Definizione delle procedure di condono».

luogo, i parametri su cui si baserà questo condono arrivano fino a prescindere dalle norme che sono state introdotte dopo il 1985, in relazione alla alla sicurezza idrogeologica. Pongo poi una domanda, alla quale vorrei avere una risposta precisa, anche in relazione all’intervento di un senatore del MoVimento 5 Stelle, che ho condiviso e voterò quegli emendamenti. Quando si parla di conferenza di servizi, scatterà il silenzio-assenso? Scatterà? Sì o no? Perché da qui partirà un meccanismo veramente inquietante. Infine, da un altro punto di vista state introducendo una disparità e una disuguaglianza tra chi ha avuto un danno

Signor Presidente, il vice presidente del Consiglio Di Maio ha detto che avrebbe chiesto la tessera del PD se lo avessimo mai ascoltato una volta parlare di condono.

Signor Presidente, quando si parla di condoni, non si parla solo di tettoie per le case al mare ma di sopraelevazioni, di case costruite negli alvei dei fiumi a rischio di esondazione e di persone che mettono a repentaglio la vita propria, dei propri figli e dei terzi: di questo si parla. (Applausi dal Gruppo PD). Avremmo immaginato che, dopo tutto quel che è accaduto, il Governo prendesse l’iniziativa di stralciare questa parte. Ha ragione il presidente Errani:

dal Gruppo PD). Qual è il patto? Che cosa si nasconde? Che cosa avete barattato per il condono edilizio? Il condono fiscale? I fanghi, di cui riparleremo? Che cosa? Dov’è questo scambio? Perché Di Maio ci tiene tanto? Vergognatevi: utilizzare la tragedia di Genova per nascondere un condono è vergognoso!

intervengo sull’ordine dei lavori. Mi è venuto un dubbio e forse qualcuno mi dovrebbe rispondere, visto che abbiamo autorevoli membri del Governo seduti in

La prima: per quale motivo l’articolo 25 si chiama «Definizione delle procedure di condono» e non ha a che fare con Genova? La seconda: io sono di cattivo carattere, Presidente, e sono andata ad aprire la Gazzetta Ufficiale

Certamente mi ricordo molto bene le tante parolacce e offese che per cinque anni abbiamo sentito dal MoVimento 5 Stelle. (Applausi dai Gruppi si è permesso, probabilmente ha preso esempio e insegnamento dal loro modo di fare. Per le parolacce mi sembra che anche in televisione, nei confronti dei giornalisti, siano i Ministri dei 5 Stelle che si dovrebbero vergognare a dirle, insolentendo giornalisti, parlamentari e

L’atteggiamento che abbiamo tenuto rispetto a questo emendamento in Commissione ha manifestato prima di tutto una profonda spaccatura all’interno della maggioranza, che si è evidenziata soprattutto nel Gruppo del MoVimento 5 Stelle, e e su cui certamente la nostra posizione politica ha agito da detonatore. Abbiamo ascoltato con molta attenzione i temi che sono stati approfonditi in discussione generale; mai come in questo caso la discussione generale è stata proficua in Commissione, ma certamente anche in Aula. Abbiamo ascoltato le voci dei territori: la caratteristica del nostro movimento politico è sempre stata quella di ascoltare con molta attenzione le voci dei territori e di non delegittimare mai, di non disconfermare mai le battaglie politiche che i nostri parlamentari hanno negli anni combattuto con impegno sui territori. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Onorevoli colleghi, ho un grandissimo rispetto di tutti gli interventi, anche profondamente critici, che sono stati fatti oggi, e anche in Commissione in questi giorni. Però non dimentichiamoci che dietro gli aridi numeri delle date anagrafiche dei condoni ci sono delle persone, delle famiglie, delle aspettative anche molto legittime, che stanno aspettando da

un approccio militaresco, che ha sempre riconosciuto e valorizzato il dissenso - prego tutti i colleghi di riconoscerci che mai e poi mai, pur assistendo ad altri atteggiamenti da parte dei colleghi di altri Gruppi parlamentari,

25.12; lo faremo coerentemente con l’atteggiamento che abbiamo tenuto qui in Aula come in Commissione. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Lo faremo e lo faremo ancora, perché noi crediamo non nell’ideologia, ma nella forza dell’applicazione vera ed attuale della nostra libertà di essere noi stessi.

Io capisco l’imbarazzo e so che vi imbarazza il termine «condono» e che cercate di usare un’altra parola. Ma proprio voi, che ci avete fatto “una capa tanta” per tutta la campagna elettorale al grido di «onestà», «legalità» e «galera» (perché la vostra ricetta è che tutto si risolve mettendo la gente in galera, meno quella che in galera ci dovrebbe andare), allora abbiate il coraggio di venire qua e di dire che avete cambiato idea. Noi idea. Noi esseri umani possiamo cambiare idea; quello che non si può fare però nelle istituzioni e in quest’Aula, è cercare di prendere per il naso noi e gli italiani.

a prendere per il naso gli italiani e a voler cambiare il linguaggio della nostra Nazione, volete il condono? Ditelo chiaramente, qua e nelle piazze. E quel bel manifesto dell’onestà e della legalità non potrete più sbandierarlo. Perché gli italiani non sono fessi: possono sbagliare, ma sono molto intelligenti nel non perseverare. Presidente, questo è l’emendamento sul quale la maggioranza ieri sera in Commissione è stata battuta. È un emendamento che noi abbiamo sostenuto perché limitava il grande messaggio che sta uscendo oggi da quest’Aula, e cioè: viva i furbi, passati, presenti e futuri. Perché è esattamente questo il messaggio che sta passando in quest’Aula. Vede, signor Presidente, ci sono cittadini italiani che per lievi difformità in questo momento sono davanti ai giudici.

Oppure, forse, diranno che ci sono cittadini italiani normali e che, invece, ci sono cittadini italiani che hanno la grazia di vivere nel collegio elettorale del vice presidente Di Maio?

solo per questo motivo cinque minuti dopo noi, dopo un appoggio che abbiamo dato a Forza Italia su questo emendamento, ci troviamo abbandonati nel voto. Ovviamente, lei capirà che questo non ci scandalizza più di tanto e non mortifica di certo le nostre convinzioni, ma, signor Presidente, certamente noi invitiamo a un ripensamento, perché vi almeno una limitazione al condono tombale che, in assenza di questo emendamento, verrebbe perpetrato.

ho già detto nell’illustrazione dell’emendamento soppressivo, voi utilizzate

in letteratura e in giurisprudenza, come il più ampio che ci sia mai stato in questo Paese. Persino i condoni successivi hanno dovuto fare i conti con le norme che nel frattempo il Parlamento aveva approvato

perché stiamo parlando soltanto delle case interessate, danneggiate o distrutte dal terremoto. Vi rendete conto che magari quelle sono proprio crollate perché erano abusive, perché realizzate dove non dovevano essere realizzate,

Cosa dobbiamo sperare? Dobbiamo sperare o altri devono sperare che arrivi un altro terremoto, un’altra calamità naturale per poter rendere sanabili le case e poter così usufruire del condono? Vi rendete conto dell’aberrazione che si sta portando avanti? Per questo vi dico: almeno questo emendamento riduce il danno. Pensateci ancora una volta perché è un’occasione per

altro che il tradimento degli elettori da parte di coloro che ieri hanno votato questo emendamento. Il tradimento lo avete compiuto voi fino in fondo. Per questo vi dico: fermatevi. Almeno su questo fronte riducete il danno.

le procedure di esame delle istanze di condono non si dovessero concludere nei sei mesi previsti. Se non dovesse succedere nulla, non si comprende che senso abbia la normativa; ben più plausibile però è l’ipotesi per cui, quantomeno in sede applicativa, si tenderà ad applicare il principio del silenzio-assenso e in tal caso questo sarebbe un gigantesco condono, visto che si tratta di pratiche giacenti da anni, un condono ad insulam. La soluzione, dunque, è quella di prevedere che, decorsi i sei mesi senza risposta, tutte le istanze si intenderanno respinte. Deve cioè essere precisato chiaramente che vale il silenzio rifiuto. A tal proposito l’ulteriore proposta è quella di estendere questo punto a tutti i Comuni d’Italia. Così facendo tra sei mesi avremo una mappa definitiva degli immobili abusivi in Italia e si potrà concretamente dare corso alla programmazione del piano straordinario di demolizioni di cui ha parlato il ministro Costa. Per queste ragioni chiedo che vengano accolti gli emendamenti a mia firma, così tra sei mesi finalmente potremo liberare l’Italia dall’abusivismo edilizio.

come modificato dalla legge n. 326 del 2003, prevede che «il rilascio del titolo abitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto». È già così.

l’assoluto vincolo per tutta l’isola di Ischia (il documento è citato all’interno di una delibera di Ischia del 17 aprile e, quindi, esiste). esiste). Che cosa succede? Ti ho fatto fare il condono, chi ha dato ha dato e chi ha avuto ha avuto. Poi basta, da qui non si fa più assolutamente niente. il concetto è che se un cittadino non ha avuto risposta nei termini del processo amministrativo può procedere all’impugnazione. In Italia è pieno di pratiche che si trascinano da anni e anni; io personalmente conosco un ente

pertanto la seguente: perché si fa tutto questo? Come è stato giustamente detto, successivamente è stato introdotto, per certe fattispecie, il silenzio-dissenso,

Sull’adeguatezza statica e strutturale degli edifici costruiti abusivamente ci sarebbe molto da dire. Dove sta il capitolato? E il diametro del tondino? La quantità di tondini? La distanza dei pilastrini? Lo spessore della soletta?

per i cittadini, per le imprese e per il territorio che è stato devastato nelle ultime settimane, dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia. Dunque proponiamo di stanziare 500 milioni di euro nel 2018 e 500 milioni di euro

quando il Parlamento europeo fu chiamato a ratificare l’Accordo sul clima di Parigi, due anni fa, ci furono 610 voti favorevoli e 38 voti contrari: tra questi 38 voti contrari figurano il voto dell’allora eurodeputato e oggi vice premier Salvini e dell’oggi ministro Fontana. Se va a parlare con i vecchi delle Dolomiti, le diranno che non hanno mai visto un evento di questo tipo, ma chi studia, chi capisce e chi non parla per niente le spiegherà che questi eventi sono collegati al mutamento ambientale e del clima.

si è stratificata, e male, nel corso del tempo. La legislazione prevede, ad esempio, che non si deve fare miscelazione di rifiuti allo scopo di diluire gli inquinanti; però si è trovato l’escamotage di collegare direttamente il sito di produzione con il sito di depurazione e, se c’è una continuità nella collettazione, non si considera rifiuto. Di fatto, quindi, la legge viene aggirata,

viene dalla depurazione di detriti industriali. Ecco come si spiega la presenza di metalli pesanti, sostanze cancerogene, oli minerali, idrocarburi pesanti, policiclici aromatici, diossine, furani e quello che volete. Prendere, anche solamente per un attimo, in considerazione il fatto che questa roba possa essere sparsa sui campi, con limiti di spargimento che sono superiori, per alcune fattispecie, al conferimento in discarica dei rifiuti pericolosi speciali, secondo me, è una follia. Anche aver inserito in tabella alcuni parametri di limitazione può essere oggettivamente non sensato. Ho contattato un tecnico di laboratorio che mi ha confermato che, per esempio, i 20 milligrammi per quanto riguarda l’arsenico sono assurdi, perché i terreni insubrici e quelli dell’agro romano contengono più di 20 milligrammi sul secco

inserire in tabella, seppure con bassi livelli, sostanze inquinanti cancerogene e persistenti come diossine e furani è un suicidio, perché la sola normativa tabellare che stabilisce dei limiti non ha senso: alcune sostanze devono essere messe al limite zero. L’operazione che dovrebbe essere fatta non è solo di revisione normativa, ma di revisione impiantistica, perché bisogna capire una volta per tutte se è tollerabile l’accumulo di metalli pesanti nel terreno, e quindi in falda, oppure no. Non ci lamentiamo se poi troviamo nell’acqua potabile parametri come arsenico, cromo e tutte queste cose. Da dove pensiamo che vengano? Vengono dalla percolazione dei fanghi sparsi. Bene aveva fatto la Regione Lombardia, che ha la competenza sui rifiuti (perché la competenza sui rifiuti è regionale), a porre un limite sugli olii minerali a 50 e bene ha fatto, ulteriormente, a vietare in 170 Comuni lo spargimento, perché si deve dare la priorità al fango zootecnico, che è privo di metalli pesanti. Chi viene a dirci che Chi viene a dirci che quelle sostanze sono fango civile, lo voglio vedere con la grattugia che gratta un po’ di acciaio inox per far uscire un po’ di cromo all’interno del refluo. Vediamo di fare un’operazione buona: questo decreto-legge scade il 28 novembre prossimo, quindi c’è tutto il tempo di mandarlo alla Camera e stralciare l’articolo 41.

La problematica principale di questi idrocarburi è il loro potenziale ecotossico e la difficoltà intrinseca a definire la tossicità a lungo termine. A questo punto, basti pensare alla presenza PFAS nella Provincia di Vicenza, che vi racconta tutto. La loro presenza non esclude la contaminazione di altri inquinanti dichiaratamente cancerogeni e mutageni con una elevata persistenza, quali metalli pesanti, diossina e IPA. La diluizione degli inquinanti ambientali sul terreno non è diversa da quella perpetrata criminalmente in tutti gli ecosistemi marini ed interrati. Ora, con questo articolo, inquiniamo per legge. Inoltre, la tossicità di questi inquinanti si aggrava quando vengono metabolizzati e bioaccumulati negli organismi lungo la piramide alimentare al cui vertice si trova inevitabilmente l’uomo, inteso come comune cittadino.

un ordine del giorno, mi pare del PD, a rivedere il tutto in prosieguo, vi inviterei a fare uno stop and go, andando a ragionare su questa tematica tanto sensibile e tanto tanto problematica, in modo da fare qualcosa di veramente serio, ma che non sia un decreto. Io mi sento offesa. A Genova ho la mia famiglia e i miei nipotini, quindi avrei votato il cosiddetto decreto Genova con tutto il cuore, per dare una mano a una città città in sofferenza. Purtroppo devo astenermi, perché non posso votare queste cose. Signor Presidente, questo articolo è l’altra ne- fandezza, l’altra vergogna nascosta dalla tragedia di Genova. si occupa di fanghi derivanti dagli impianti di depurazione: impianti di depurazione - cito testualmente - delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili o da insediamenti civili e produttivi o anche provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi; quindi, anche da acque reflue derivanti da industrie. Non è vero, signor sottosegretario Crimi, che si è andata a sanare una questione irrisolta e non regolata da anni. Con questo articolo non fate altro che far riferimento al decreto legislativo n. 99 del 1992,

fate l’eccezione per gli idrocarburi? Perché ritenete di poter elevare le soglie di presenza di tali sostanze nei fanghi che vanno sui nostri terreni, dove si coltivano

Avete fatto eccezioni anche per il cromo, l’arsenico, il selenio, il toluene. Perché avete l’esigenza di far sì che queste sostanze nocive possano essere maggiormente presenti nei fanghi? Ecco perché - e concludo - non solo insistiamo sulla soppressione di questo articolo vergognoso, ma voteremo anche gli altri emendamenti presentati dal collega De Bonis della mia Regione. È certo, e ripeto della mia Regione, perché aumentare la soglia degli idrocarburi nei fanghi significa rovinare soprattutto persone che vivono nelle Regioni dove si fanno le estrazioni petrolifere. Eppure, solo nella scorsa legislatura vi eravate dipinti le mani. Non ci facevate votare. Da quel banco non potevamo accedere sullo sblocca Italia perché dicevate che stavamo avvelenando. Voi state avvelenando con questo articolo. Avete già svenduto tutto. Siete passati dall’essere ambientalisti - come ha ben detto prima la collega - addirittura al fatto gli idrocarburi, il cromo e l’arsenico dei fanghi di depurazione. Siamo veramente impazziti! E poi vi permettete di chiamare traditori colleghi seri, autonomi e liberi, che non fanno nient’altro che continuare a dire le cose che dicevate cinque anni fa!

contro la libertà e contro l’autonomia delle persone. Prima o poi si va a sbattere. E noi vi aspettiamo, perché sbatterete.

raccolgo le preoccupazioni che sono emerse nel dibattito e prendo anche atto della necessità di una revisione della norma intera che riguarda, appunto, la questione dei fanghi di depurazione.

hanno gli impianti depurazione e da sempre, fino all’entrata in vigore di una sentenza del Tar della Lombardia, hanno distribuito i fanghi in agricoltura, con tutta una serie di limiti e questioni precise che non andavano nella direzione di essere contro la salute del cittadino. No anzi, tutt’altro. Si è colta - credo l’occasione

il quale l’articolo 41 ha posto un limite allo spargimento dei fanghi; quel limite che era stato stabilito da un giudice con la sentenza del TAR Lombardia. Mi sarei aspettata dal Governo una maggiore una maggiore incisività sul carattere transitorio di questa norma che - come sappiamo - gestisce un’emergenza. Dietro al tema dei fanghi sappiamo esserci problemi di tutela ambientale, di tutela della salute, ma anche problemi di sostenibilità economica, quelli ai quali faceva riferimento

dice che dalla depurazione delle acque possono derivare fanghi dai quali si può estrarre il fosforo, che è una sostanza estremamente importante in agricoltura, e sappiamo che nei prossimi dieci anni potrebbe andare in esaurimento. La invito, Sottosegretario, a vedere che cosa stanno facendo altri Paesi, come Svizzera